i prodotti che dal maiale derivano, i prosciutti che ci hanno resi famosi in tutto il mondo, rischiano uno stop delle importazioni. Già il Canada ha chiuso le frontiere, come il Giappone e la Thailandia. Rischiamo il mercato degli Stati Uniti. Rischiamo quindi una tragedia. c'era stato incontro tra il commissario e le parti interessate, gli agricoltori e i trasformatori. Purtroppo, le date che il commissario aveva dato, relative al provvedimento che sarebbe stato adottato dall'Unione europea, non sono state rispettate, perché tutto è stato anticipato di qualche giorno e questo determina che la messa in sicurezza dei maiali sarà di fatto impedita. Per questi motivi noi chiediamo al Governo e in particolare al ministro Lollobrigida di venire in Aula e riferire

dello scorso anno. Non ci voleva che nella Food Valley, famosa in tutto il mondo per la qualità del suo cibo, ci fosse una tragedia così imminente. Sono due anni che la peste suina dovrebbe essere debellata in modo efficace e si fanno solo chiacchiere. Capisco l'importanza di leggi come il premio del cuoco e i giovani in agricoltura, gli agricoltori sentinelle del territorio, ma poi, quando si presentano problemi forse bisognerebbe avere risposte più efficaci e solerti.

onorevoli senatori, il prossimo 28 luglio il Venezuela sarà chiamato al voto per le elezioni presidenziali, a distanza di sei anni dalle elezioni che, boicottate dall'opposizione, segnate da un forte astensionismo e ritenute non credibili da larga parte della comunità internazionale, avevano portato al rinnovo del mandato presidenziale per Nicolas Maduro. Dopo una stagione politica ed economica drammatica - segnata da gravi conseguenze sul piano sociale, da sistematici episodi di violenza da parte delle autorità governative, dall'incertezza del quadro giuridico, dall'inaffidabilità del sistema giudiziario, dall'arbitrarietà dell'azione amministrativa, dal crollo degli investimenti stranieri, dalla drastica contrazione del prodotto nazionale lordo e dalla crescita esponenziale dei livelli di povertà della popolazione dal mese di agosto 2021, di un processo negoziale tra il regime venezuelano e la Piattaforma unitaria democratica, l'organismo che riunisce le principali anime dell'opposizione democratica, in vista dell'organizzazione nel 2024 di elezioni presidenziali libere, eque ed inclusive e della revoca delle sanzioni economiche che gravano da anni sul Paese, aveva lasciato intravedere la possibilità che in Venezuela potesse avviarsi verso un periodo di riconciliazione e di democratizzazione. Il traguardo più importante di questa stagione di dialogo è stata la sottoscrizione, il 17 ottobre 2023, nello Stato caraibico di Barbados, di due accordi parziali sulla promozione dei diritti politici e delle garanzie elettorali per tutti e sulla protezione degli interessi vitali della Nazione, con l'impegno allo svolgimento di elezioni presidenziali libere ed inclusive nella seconda metà del 2024, previo aggiornamento delle liste elettorali, anche all'estero, da tenersi alla presenza di missioni internazionali di monitoraggio elettorale. Dopo che il 22 ottobre 2023 le primarie organizzate dalle forze di opposizione, cui hanno partecipato oltre 2 milioni di cittadini, hanno visto prevalere nettamente Maria Corina Machado, la *leader* del partito Vente Venezuela, quale possibile candidata unitaria di tutte le opposizioni in vista delle elezioni presidenziali, l'azione repressiva posta in essere dal regime venezuelano è stata riattivata. La stessa Maria Machado, già sanzionata con misure restrittive dieci anni fa, è stata nuovamente colpita da un provvedimento di ineleggibilità nel gennaio 2024, mentre ulteriori interdizioni ai candidati sono state irrogate a danno di altre personalità politiche di rilievo nella scena politica venezuelana. Alla fine del mese di gennaio 2024, la stessa Corte suprema del Venezuela ha respinto il ricorso di Maria Corina Machado in merito all'interdizione ad ogni carica pubblica inflitta a suo carico, con una pronuncia che rende incerto il percorso di riconciliazione e democratizzazione del Paese. Come ha ricordato la stessa Maria Corina Machado, audita lo scorso 30 gennaio della 3a Commissione permanente del Senato, appare assolutamente necessario che in vista delle elezioni presidenziali, tutti i venezuelani siano messi in condizione di votare, anche quelli residenti all'estero, e che venga assicurata protezione internazionale agli attivisti politici che lavorano nel Paese. Tenuto conto che la crisi interna venezuelana ha delle fortissime ricadute anche sul piano regionale e internazionale, contribuendo ad alimentare focolai di tensione e di instabilità politica che rischiano di avere effetti ulteriormente destabilizzanti per gli interi equilibri del Continente americano, e che la stabilità democratica e il ripristino di indifferibili condizioni di sicurezza e di legalità in Venezuela sono indispensabili, al fine di tutelare l'incolumità dei cittadini appartenenti ai membri della numerosa comunità italo-venezuelana presente nel Paese, la Commissione affari esteri e difesa del Senato ha ritenuto necessario prendere posizione in modo significativo sulla questione. Con la presente risoluzione, votata - ci tengo a dirlo - all'unanimità della Commissione affari esteri e difesa del Senato, nella convinzione che lo svolgimento di elezioni libere e regolari rappresenti una condizione irrinunciabile dei Paesi democratici e che l'organizzazione di processi elettorali indipendenti e trasparenti sia indispensabile per promuovere un ambiente elettorale competitivo e la fiducia dei cittadini e l'integrità delle elezioni e delle stesse istituzioni democratiche, si impegna il Governo italiano: a ribadire in ogni consesso internazionale l'importanza del ripristino della democrazia, dello Stato di diritto e del libero esercizio dei diritti civili e politici da parte della popolazione del Venezuela, richiamando le autorità di Caracas alla necessità di rilasciare i prigionieri politici, e far cessare ogni azione volta a impedire una reale partecipazione democratica alle prossime competizioni elettorali; ad intraprendere ogni iniziativa utile ai fini dell'attuazione degli Accordi di Barbados, con particolare riguardo alla definizione di un cronoprogramma, all'aggiornamento del registro degli elettori, anche all'estero, e all'autorizzazione alla presenza di missioni internazionali colleghi per cortesia a sostenere l'azione diplomatica dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri, finalizzata a definire una posizione comune dei 27 Paesi dell'Unione sulla linea del presente atto d'indirizzo; intraprendere ogni iniziativa utile a livello diplomatico nelle sedi internazionali affinché le elezioni presidenziali previste nella seconda metà del 2024 in Venezuela siano libere, eque, inclusive e credibili e e si svolgano in modo trasparente, consentendo anche ai legittimi rappresentanti dell'opposizione di prendervi parte in qualità di candidati; a esperire ogni ulteriore azione utile a tutelare la comunità italiana in Venezuela e le aziende italiane tuttora operanti in quel Paese e i loro legittimi interessi economici. Dopodiché, signora Presidente, chiedo di apportare una modifica al quinto impegno della bozza di risoluzione in esame: in occasione dell'approvazione in Commissione, non conoscendo ancora la data delle elezioni, si era scritto «nella seconda metà del 2024», come ho letto; ora sappiamo che il Presidente del Consiglio nazionale elettorale in Venezuela ha indetto le elezioni presidenziali per il 28 luglio 2024. PRESIDENTE. Quindi aggiungiamo la data? CRAXI

e li ha costretti a esodi biblici verso i Paesi confinanti. Il regime di Maduro è sostenuto soltanto dai peggiori Stati canaglia di tutto il mondo e questa non può che essere la premessa rispetto a qualsiasi discussione che apriamo sul Venezuela. Mi lasci dire allora,

la volontà dell'Unione europea di riconoscere la Presidenza costituzionalmente prevista dell'allora presidente del Parlamento venezuelano Juan Guaidó.

possiamo dire che il Presidente eletto mancava, perché il presidente Maduro era stato eletto con elezioni truffaldine fraudolente, riconosciute come tali da tutti, a partire, tra l'altro, dall'allora ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi. Milanesi. Tra le altre cose, noi non abbiamo ancora un ambasciatore, ma siamo rappresentati da un incaricato d'affari. Ma ciò non fu sufficiente a prendere la posizione che avremmo dovuto prendere e che tra l'altro la resistenza anti-chavista venezuelana ci chiedeva di prendere; una posizione chiara che ci distinguesse dall'Iran, dalla Cina, dalla Corea del Nord e da Paesi di questo stampo. L'Italia non lo fece, secondo me voltando le spalle a un Paese che, nel suo stesso nome, denuncia il legame di sangue che intercorre con il nostro Paese. Venezuela vuol dire "piccola Venezia"; è un Paese che già con la sua stessa denominazione ci ricorda quanto sangue italiano, quanta carne, quanta vita italiana ci sia lì. Ebbene, noi

l'indimenticato presidente della Commissione affari esteri del Senato Petrocelli o l'altrettanto indimenticato - ahinoi - sottosegretario per gli affari esteri Manlio Di Stefano, che erano addirittura andati in Venezuela a fare una visita e che tornarono dicendo che i corsi di educazione musicale che si tenevano in Venezuela erano di primario livello, per non parlare poi del sistema elettorale che il Venezuela aveva adottato. Ecco, di questo si parlava, di un affare interno del Venezuela, mentre l'allora ministro dello sviluppo economico e del lavoro, nonché vice presidente del Consiglio dei ministri, Luigi Di Maio andava a trovare i gilet gialli in Francia, che mettevano a ferro e fuoco il Paese, provocando anche dei morti. Quello non era un affare interno della Francia; lì si poteva andare, senza neanche avvisare il Governo in carica. Ecco, c'era questa divisione.

lucidità politica e di maggiore dignità a livello internazionale per il nostro Paese, che io credo sia ben rappresentato da questa risoluzione. Una risoluzione che interviene in un momento nel quale, tra le altre cose, il Venezuela crea problemi anche di politica estera nella regione dell'America del Sud, nel senso che appunto Maduro non si

Voglio sempre ricordare e ringraziare l'indefesso lavoro del presidente Casini, che è qui in Aula, che è stato determinante per risolvere alcune crisi e per mettere a disposizione la nostra rappresentanza diplomatica, salvando letteralmente la vita a dissidenti del regime. Ebbene, il Governo di Maduro, come sapete, sta avanzando addirittura rivendicazioni territoriali nei confronti di Paesi vicini: vorrebbe prendersi un pezzo della Guiana, come se nulla fosse, e vorrebbe della Guiana, come se nulla fosse, e vorrebbe portarlo via con un colpo di matita sulle mappe geografiche. C'è un problema grosso aperto con il Cile di Gabriel Boric, dove sono stati consumati degli omicidi a sfondo politico che il Governo cileno ha abbastanza apertamente addebitato a dei mandanti politici che stanno seduti a Caracas.

di candidare una figura nobile, una donna riconosciuta *super partes*, come Corina Yoris; sostanzialmente anche questo tentativo sta andando a vuoto. Dunque è importantissimo che

il dovere storico, culturale e politico di essere presenti in quella fase. Dal canto nostro, c'è il massimo sostegno al Governo perché inverta la rotta del 2018 e faccia sentire stentorea e forte la propria voce, anche a riconferma dei nostri legami con la comunità italiana venezuelana, con i milioni di venezuelani di origine italiana, che magari non hanno un passaporto, ma che ancora sentono forte il legame con chiamare la madrepatria, e perché faccia sentire anche la nostra presenza a tutela dei diritti democratici e delle libertà. L'Italia non può stare da nessun'altra parte che da quella e credo che ogni posizione che non sia fermamente dalla parte dei diritti democratici e delle libertà sia una posizione contro i diritti democratici e le libertà. Non c'è una possibilità terzista: o si sta dalla parte della libertà o si sta dalla parte della tirannia; o si sta dalla parte della democrazia o si sta dalla parte della dittatura. Il nostro Paese, la nostra Costituzione, la nostra storia, la nostra tradizione politica ci impongono di essere da quella parte. Quindi è apprezzabile che il Parlamento dia un mandato forte al Governo italiano e all'Unione europea, perché prendano una posizione e pretendano una transizione democratica in Venezuela.

economica, ma anche politica, sociale e democratica. A dieci anni dall'insediamento di Maduro e a venticinque dalla presa del potere del suo ispiratore Hugo Chavez, quello che era uno degli Stati più ricchi e solidi dell'America Latina presenta indici di povertà e disoccupazione altissimi, un'inflazione fuori controllo e un tasso di delinquenza e corruzione fra i più alti al mondo. alcuni numeri che fotografano la situazione: più del 90 per cento dei venezuelani vive sotto la soglia della povertà; in alcuni anni l'inflazione in Venezuela si è attestata tra il 150 e il 400 oltre 7 milioni di venezuelani hanno lasciato il Paese e Caracas è stata classificata come la città più violenta al mondo. Questa crisi umanitaria è tra le peggiori del millennio, insieme a Siria, Afghanistan e Ucraina. Incapace di affrontare la situazione con gli strumenti democratici, Chavez prima e Maduro oggi hanno poco a poco compresso ogni libertà, hanno arrestato i propri oppositori e hanno falsato la competizione democratica con elezioni farsa o dichiarando ineleggibili i più pericolosi rivali politici. Negli ultimi dieci anni oltre 15.000 persone sono state arrestate per motivi politici. In poche parole, tutte le garanzie dello Stato di diritto sono state calpestate pur di permettere alla cricca al potere di sopravvivere. Un potere che si regge ormai sull'uso della forza, la corruzione e l'assoggettamento dei media, della magistratura e, soprattutto, dei militari. La parabola del *chavismo* contiene molti insegnamenti e parla anche a noi occidentali, in particolare a noi europei. Essa, infatti, rappresenta la sconfessione pratica di quell'ideologia che, presentandosi come il socialismo del ventunesimo ha affascinato non pochi intellettuali occidentali, sempre pronti ad appoggiare qualsiasi ideologia si presenti come critica dei nostri valori e del nostro sistema politico. Intellettuali che spesso, ancora oggi in preda ad uno strabismo strano, non riescono a chiamare con il suo nome la dittatura di Maduro o semplicemente voltano lo sguardo dall'altra parte quando sentono parlare dei suoi misfatti. È stato proprio il tentativo di nazionalizzare le enormi risorse petrolifere di cui è ricco il Paese, di combattere la proprietà privata ed il profitto imprenditoriale e di controllare i prezzi, in una parola di imporre dall'alto uno statalismo statale assoluto, che ha portato il Venezuela allo stato attuale, mostrando a tutti che quell'ideologia, sconfitta più volte dalla storia, è sempre uguale a se stessa nel portare povertà e comprimere la libertà umana. Con questa risoluzione, consapevoli delle difficoltà in cui versa il popolo venezuelano, intendiamo richiamare il Governo, l'Europa e tutto il mondo libero a impegnarsi con rigore e incisività nei consessi internazionali per far rispettare dal Governo venezuelano gli impegni presi. In particolare, Maduro dovrà garantire che le prossime elezioni presidenziali si svolgano in piena libertà e trasparenza e che tutti i partiti dell'opposizione democratica saranno messi in condizione di concorrere e contendersi la *leadership*. Necessario, altresì, l'immediato rilascio dei tanti oppositori politici incarcerati senza giudizio o senza un giusto processo. Un appello particolare lo rivolgiamo al nostro Governo, nella consapevolezza che antichi e forti rapporti legano i nostri due popoli, testimoniati fra l'altro dalla presenza massiccia in Venezuela di cittadini di origine italiana. Nel Paese latino-americano, l'Italia ha poi ancora oggi interessi commerciali ed economici che vanno difesi e tutelati, a cominciare da quelli delle tante nostre aziende che vi operano e commerciano. Difendere la libertà, anche in un Paese geograficamente lontano, non è né inutile, né poco importante. Significa, infatti, difendere anche la nostra libertà. Questa risoluzione, pertanto, è un invito ad essere più incisivi ed efficaci, facendo valere tutte le armi diplomatiche e politiche a nostra disposizione.

signor Presidente, desidero ribadire a quest'Assemblea come l'Italia e quindi il Governo seguano con attenzione la crisi del Venezuela e auspichino che il Governo di Maduro ponga in essere quanto stabilito dagli accordi di Barbados tra Esecutivo e opposizione lo scorso ottobre. Ci aspettiamo che venga garantito lo svolgimento di elezioni presidenziali libere ed inclusive a luglio, secondo il calendario costituzionale. Seguiamo con attenzione l'evolversi della campagna elettorale in Venezuela e auspichiamo il rispetto di tutte le norme democratiche, del pluralismo e dello Stato di diritto. All'opposizione devono essere riconosciuti diritti civili e spazio democratico. In base agli accordi di Barbados ci aspettiamo che le autorità venezuelane consentano il pieno svolgimento delle missioni internazionali di monitoraggio elettorale, tra cui quella dell'Unione europea. Ricordo a quest'Aula gli ultimi sviluppi negativi avvenuti nel Paese: il mancato riconoscimento del risultato delle primarie dell'opposizione, l'arresto dell'attivista *Rocio* San Miguel, la decisione del Governo di Caracas di sospendere l'attività dell'Alto Commissario Onu per i diritti umani, i continui atti ostili verso le opposizioni, da ultimo con i mandati d'arresto annunciati dal Governo a marzo, alcuni dei quali nei confronti dei cittadini italo-venezuelani. Ci aspettiamo, come Governo, un'immediata ripresa delle attività dell'Alto commissario per i diritti umani, con il rientro in Venezuela dei funzionari ONU espulsi dal Paese. Monitoriamo la questione dei prigionieri politici ancora in carcere, tra cui purtroppo tanti cittadini italiani, dei quali continuiamo a richiedere in ogni occasione il rilascio. In particolare, stiamo seguendo casi dei concittadini Juan Carlos Marrufo e Alfredo Oreste Schiavo, date le loro precarie condizioni di salute. Così come seguiamo con preoccupazione gli sviluppi della disputa tra Venezuela e Guyana in merito alla regione dell'Esequiba. Riteniamo che la questione vada ricondotta nell'alveo del diritto internazionale. Infine, tramite l'azione del nostro incaricato d'affari in Venezuela e console generale a Caracas, stiamo lavorando per garantire ogni tutela alla numerosa collettività italiana presente nel Paese.

Signora Presidente, innanzitutto sottopongo una questione tecnica. Preliminarmente, vorrei chiedere alla Presidenza di segnalare agli Uffici di poter apporre anche la firma di chi le parla alla risoluzione, perché, per un problema esclusivamente di natura tecnica

solo apparentemente, a fronte di un'analisi superficiale e distratta, come troppe volte si compie, talvolta anche in quest'Aula, certamente negli spazi della formazione della pubblica opinione, sui mezzi di comunicazione e nel dibattito nella nostra società civile, società civile, può sembrare lontana, distante, non interessante per i nostri destini e la nostra collettività. In realtà, il tema del Venezuela è una gemma di una corona, la corona dalla storia, che stiamo attraversando. Noi dobbiamo avere la piena consapevolezza che quello che oggi accade in un Paese che sembra così distante, ma che in realtà sia per gli aspetti di natura culturale, storica e identitaria, cui giustamente ha fatto riferimento nel suo intervento il collega senatore Scalfarotto, sia per gli assetti geopolitici, è una questione che ci riguarda. è una questione che ci riguarda. Ci riguarda innanzitutto dal punto di vista delle questioni di fondo etico-valoriali: il tema della difesa dei diritti umani, della tutela delle libertà, della salvaguardia delle prerogative che noi riteniamo essere universali, come la libertà di parola, il diritto di cittadinanza, l'espressione di voto, la libera stampa, tutte questioni che noi riteniamo essenziali e fondamentali. Pertanto, avendo noi subito nella nostra storia chi ha voluto conculcare, limitare, deprivare questo tipo di libertà, abbiamo il dovere morale

poi un secondo aspetto, parallelo rispetto a ciò, che tiene in considerazione che cosa rappresenta un Paese come questo sullo scacchiere complessivo ed internazionale e il peso, la rilevanza, l'interessenza delle politiche compiute dal Venezuela, che possono influenzare, se non addirittura determinare, una serie di scelte che, in maniera diretta o indotta, possono anche arrivare all'interno delle nostre comunità. Discutere di questa tematica non è quindi discutere di una questione astratta: significa discutere di questioni che attengono direttamente al nostro sistema valoriale, alla nostra collocazione in politica estera e nel sistema delle relazioni internazionali. E dico ciò anche perché - e qui vengo al merito della questione non vi è chi non veda che il Venezuela è un pezzo di quella tensione destinata purtroppo ad attraversare il secolo attuale. Così come il secolo breve, il Novecento, è stato caratterizzato dalla tensione, dallo scontro in alcuni casi anche dalla guerra (prima calda e cruenta e, poi, fredda) fra il sistema delle liberal-democrazie e i sistemi totalitari di destra e di sinistra, dei nazi-fascismi e dei comunismi reali, noi rischiamo che quello attuale sia il secolo della tensione, e in alcuni casi è già della guerra, che speriamo non si allarghi. Il nostro compito deve essere quello di suturare queste ferite, che si stanno pericolosamente allargando, fra il sistema delle liberal-democrazie, da un lato, e il sistema delle autocrazie, dall'altro. Perché il Venezuela si inserisce all'interno di questa cornice? cornice? Noi dobbiamo avere la consapevolezza di guardare dal punto di vista complessivo la vicenda. Non possiamo limitarci a ragionare puntualmente sui singoli momenti di sfrido che arrivano quasi quotidianamente alla nostra discussione se perdiamo di vista la logica d'insieme. Dentro questi punti di sfrido stiamo oggi conoscendo vicende drammatiche perché l'Ucraina, il Medio Oriente e il Mar Rosso sono le tre faglie di Sant'Andrea sulle quali i due blocchi delle liberal-democrazie - da un lato - e delle autocrazie - dall'altro - scorrono, si toccano e sprigionano l'energia che determina purtroppo tensione, guerra e morte. Noi sappiamo che c'è un ulteriore momento di sfrido, che oggi è congelato e che la capacità della politica deve mantenere in termini di attuale situazione di *status quo,* che si chiama Taiwan. Non voglia il cielo che anche da quel versante si riapra una tensione di carattere bellico che rischierebbe di innescare situazioni non più recuperabili. Il Sud America è all'interno di questo tema di carattere globale e non possiamo pensare che sia una monade. Dice qualcosa il fatto che oggi il Venezuela è il luogo nel quale gli Hezbollah - sì, gli Hezbollah sono un pezzo dell'economia illegale del Paese, costruiscono e costituiscono una serie di legami con i cartelli e realizzano attività illegali connesse alla produzione e al commercio illegale di droga di stupefacenti sul piano globale? Ci dice qualcosa questo elemento? Ci dice qualcosa che Iran e Venezuela, due Stati paria, sono legati intimamente da relazioni diplomatiche, amicizie politiche e collaborazioni militari? Perché tutto questo avviene? Avviene evidentemente nel quadro di una strategia globale. La presenza in questi termini di una realtà che si può configurare, o che taluni richiedono anche di configurare al rango di un'organizzazione terroristica - peraltro presente non soltanto in Venezuela, ma anche in Nicaragua - ha degli obiettivi molto precisi: molto precisi: diminuire lo svantaggio geografico che c'è fra il comparto dell'Est (Russia, Cina e Iran) e quello dell'Ovest e creare una spina nel fianco degli Stati Uniti d'America. Più in generale, ha l'obiettivo di tentare di rompere il principio della dottrina Monroe, sulla quale gli Stati Uniti d'America hanno costruito tutta la loro politica estera da che

e dell'ascolto soltanto delle ragioni di chi è sul campo, quasi come se fossimo il sensale del mercato che poi prova a trovare un punto di convergenza occasionale, se non conveniente. *(Applausi)*. Non è così che si fa politica estera. La politica estera si fa sapendo di essere coerenti nel quadro del sistema dei valori ai quali si è ancorati. E mi permetta di dirlo, signora Presidente, nella settimana in cui (e concludo) il nostro Presidente della Repubblica, che ancora ringraziamo, ha pronunciato, in occasione della celebrazione dei settantacinque anni della NATO, parole molto precise, molto chiare e illuminanti su cosa significa stare all'interno delle organizzazioni internazionali in coerenza con il nostro dettato costituzionale, sapendo che attraverso questo esercizio nascono l'interesse nazionale e la nostra capacità di essere un Paese realmente all'altezza delle sfide della storia. È per questo che la risoluzione al nostro esame è importante. È per questo che il Venezuela non è una monade. È per questo che noi abbiamo il dovere di approvarla.

Il risultato elettorale determinerà anche il Governo del Paese sudamericano per i prossimi sei anni. La risoluzione della Commissione affari esteri chiede quindi di garantire lo Stato di diritto, il pluralismo, la democrazia, il controllo internazionale sulla regolarità del voto: cioè reclama che le elezioni si svolgano in un clima di pieno e sereno confronto con i candidati dell'opposizione democratica e vi sia quindi la più ampia partecipazione popolare. Va ricordato che Nicolas Maduro è al potere dal 2013, cioè da undici anni, dopo aver vinto anche le elezioni presidenziali del 2018, considerate però irregolari e non riconosciute dall'ONU e dall'Unione europea, dove ha votato meno della metà degli aventi diritto. Ovviamente sta lavorando attraverso gigantesche pressioni sull'opinione pubblica e una propaganda sfrenata che punta alla propria rielezione, con campagne pubblicitarie in suo favore, che coinvolgono tutti i media. Super Baffo è persino il titolo di un cartone che magnifica le gesta di un supereroe che - guarda caso - sembra proprio Maduro, che vuole raggiungere un consenso sempre più ampio. Va ricordato altresì che il partito di Maduro ha perso le elezioni parlamentari nel 2015, gestendo il potere in un periodo di cosiddetta "anatra zoppa" e un'Assemblea nazionale con una maggioranza allineata all'unità nazionale, che non corrispondeva al suo schieramento, il grande polo patriottico, che poi è tornato, nel 2020, a vincere le elezioni dell'unica Camera venezuelana. La risoluzione della Commissione affari esteri chiede che chiunque voglia possa esprimere il proprio voto, inclusa la vasta comunità di diverse migliaia di cittadini venezuelani residenti in Italia, e che il voto sia libero, democratico e trasparente. Va ricordato che i legami tra l'Italia e il Venezuela sono sempre stati storicamente molto vasti e articolati, posto che la comunità italiana in Venezuela conta 160.000 nostri connazionali registrati nei due consolati, Caracas e Maracaibo, su un totale di più di circa 26 milioni di abitanti. Non si Non si può dire altrettanto dei rapporti attuali, che hanno visto ridurre soprattutto le reciproche relazioni commerciali, posto che il Venezuela è un Paese sottoposto a una serie di sanzioni internazionali e molti Paesi, inclusa ovviamente l'Italia, hanno limitato o interrotto molti dei propri investimenti. Gli indici di rischio sono molto alti per chi voglia investire, nonostante si tratti di un Paese con grandi potenzialità, ancora in larga parte da sviluppare e costruire, che inoltre dispone di una grande ricchezza di risorse naturali e materie prime. Va ricordato che il Venezuela è tra i membri fondatori membri fondatori dell'OPEC, l'organizzazione degli esportatori di petrolio, e possiede una delle più ampie e vaste riserve di greggio al mondo. Anche a causa delle sanzioni in atto, non è più tra i maggiori produttori di oro nero. Questo incide ovviamente sull'economia e sul prodotto interno lordo, che è crollato dagli oltre 400 miliardi di dollari del 2014 ai poco più di 40 stimati nel 2020. Il petrolio, peraltro, è stato uno dei punti di forza del regime di Chávez fino al 2013, facendone uno dei principali esportatori. Eppure la volontà di uscire da anni di recessione e di aprire agli investimenti internazionali ha fatto registrare, proprio negli ultimi anni, un aumento di investimenti esteri, soprattutto da parte di Paesi come Cina, Russia e Turchia, e una crescita dell'economia grazie alle agevolazioni, alle società private e a un sistema fiscale molto attraente, che ha riportato il PIL a oltre 100 miliardi nell'ultimo anno. Ha contribuito alla crescita anche l'alleggerimento delle sanzioni statunitensi, dopo l'apertura di un processo democratico ai principali partiti di opposizione. Ma le sanzioni statunitensi potrebbero tornare in caso di una nuova involuzione democratica. Quindi è necessario tenere alta l'attenzione alle pressioni internazionali. La crescita economica ha avuto un impatto positivo per moderare l'inflazione, ancora molto alta, e sostenere il potere di acquisto dei venezuelani, dove permane un forte livello di disoccupazione. Ecco quindi che Maduro, malgrado tutto, si presenta alle elezioni con risultati misurabili, nonostante le sanzioni internazionali e l'ostilità della comunità internazionale, dovuta all'evidente compressione dei diritti e alla limitazione dei processi democratici. Detto questo, noi auspichiamo che in Venezuela, dove al momento sembra assicurata la presenza di più candidati a presidente, si possano tenere elezioni presidenziali libere e democratiche. Auspichiamo che il Paese sudamericano possa ritrovare la piena libertà e i fasti di un tempo, come merita. Ne vanno anche dell'interesse e della stabilità dell'intera regione e degli equilibri internazionali. Pertanto annuncio il sostegno convinto e il voto favorevole dei senatori di Forza Italia alla risoluzione che chiede maggiore democrazia e maggiore trasparenza nelle prossime elezioni, assieme alla richiesta di garanzie di tutela degli interessi italiani e delle aziende italiane in Venezuela. *(Applausi)*.

Non è un ringraziamento di rito, presidente Craxi, ma è una cosa sentita. È raro vedere la Commissione unita, esprimere un'unità di intenti e riportarla in Aula in questo modo. Quindi, ringrazio anche i Gruppi politici che hanno partecipato alla stesura Ricordo che l'iniziativa è nata subito dopo la videoconferenza che abbiamo tenuto in Commissione esteri, a fine gennaio, con la

difficilissimo farla dopo i fatti che lei aveva esposto. Ricordo che la sensazione fu quella di impotenza, direi di incredulità: com'è possibile che succeda ancora al mondo una cosa del genere. Subito dopo l'audizione in Commissione sono andato a rivedermi gli atti e i documenti che Amnesty International e Foro Penal hanno pubblicato dal 2018 in poi, che parlavano di bambini detenuti, oppositori detenuti ingiustamente, civili processati in tribunali militari; 3 milioni di sfollati, 3 milioni di persone scappati dal Venezuela per rifugiarsi negli Stati vicini; una folta comunità di italiani in Venezuela in difficoltà. Era impossibile da parte nostra far finta di niente - come qualcuno ci ha accusato poco tempo fa - ho ritenuto che fosse non utile, ma decisamente importante, apporre la mia firma e la firma del Gruppo del MoVimento 5 Stelle a questa iniziativa. Ricordo anche che a ottobre ci fu uno spiraglio di luce in quanto gli accordi di Barbados lasciavano intravedere una possibile soluzione. In cambio di una piccola concessione al regime di Maduro, riguardo le sanzioni che attualmente vigono contro il suo Paese, si impegnava il regime a garantire elezioni libere al popolo venezuelano e a permettere agli oppositori di presentare un proprio candidato. Bene: pochissimi giorni fa, il regime di Maduro ha arrestato altri sette membri dello *staff* di Maria Corina Machado. Sta costantemente cercando di eliminare ogni oppositore e di impedire che vi sia un concorrente per le elezioni presidenziali. Credo che questo non sia ammissibile.

oltre alle sanzioni già in essere - a cambiare idea, per permettere finalmente al popolo venezuelano, di cui c'è una rappresentanza qua in Aula, di esprimere un Governo che lo rappresenti. L'impegno di ribadire in ogni consesso internazionale l'importanza del ripristino della democrazia mi sembra quindi un punto assolutamente da portare avanti; intraprendere ogni iniziativa affinché il Governo di Maduro rispetto agli accordi di Barbados, che ha sottoscritto. Quindi, va assolutamente perseguito questo secondo impegno, di adoperarsi affinché i numerosi cittadini venezuelani residenti in Italia possano votare. Come si fa a non sottoscrivere un impegno di questo tipo?

l'impegno a esperire ogni azione utile a tutelare la comunità italiana in Venezuela: credo che questo sia un percorso da intraprendere con forza dal Governo, che ci troverà ovviamente al suo fianco affinché tutto

Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, la prima elezione alla Presidenza del Venezuela di Nicolas Maduro nel 2013 ha sancito l'inizio di un periodo notoriamente caratterizzato da un regime autoritario alquanto poliziesco, che sembra aver portato il Paese verso la perdita dei valori democratici. Sintomo della perdita di quegli *standard* democratici essenziali è stato che, da quel momento in poi, le tornate elettorali successive hanno visto un forte astensionismo da parte della popolazione. Tutto ciò risulta al giorno d'oggi inconcepibile in uno Stato come il Venezuela, che da sempre intrattiene rapporti privilegiati con il mondo occidentale, per questioni legate non solo ad affinità storiche, culturali e sociali, ma anche a un solido interscambio economico. Proprio per questi motivi, alle prossime elezioni presidenziali venezuelane di quest'anno sarà fondamentale fare tutto ciò che è in nostro potere perché siano libere, trasparenti e pluraliste, promuovendo l'integrità delle istituzioni democratiche e dei processi elettorali, nel rispetto della fiducia dei cittadini. Per perseguire lo scopo di veicolare le elezioni dall'interno e per permettere al regime di Maduro di riaffermarsi negli anni successivi alla sua prima Presidenza, si è assistito a una sistematica violazione dei diritti umani in Venezuela. Venezuela. Le stesse Nazioni Unite hanno rilevato una serie di crimini contro l'umanità commessi da esponenti del Governo di Maduro: giornalisti, oppositori politici e attivisti sono sistematicamente imprigionati, interdetti da cariche politiche e privati di ogni esercizio di libertà e diritto di espressione che non sia conforme al regime. Questa è evidentemente una violazione dei diritti dei cittadini, una privazione della loro libertà decisionale, che si traduce in una retrogressione nel cammino democratico del Paese. È per queste ragioni che le elezioni del 2024 potrebbero rappresentare un punto fondamentale verso il ritorno alla democrazia. Ma, perché sia così, è necessario intervenire in termini diplomatici per favorire il ritorno verso la strada democratica del Venezuela. Basti pensare all'attivista per i diritti umani ed ex candidata Maria Machado, che abbiamo avuto l'onore di vedere in audizione lo scorso gennaio presso la Commissione affari esteri e difesa, a cui in tutti i modi è stato impedito di candidarsi alle elezioni politiche in opposizione a Maduro, solo perché alle primarie aveva conquistato una cospicua parte di elettorato e avrebbe potuto rappresentare una seria minaccia per il regime. Questo è quanto che generalmente succede nei regimi dittatoriali; al contrario, tutto ciò è impensabile se applicato a un contesto che vorrebbe essere democratico, come quello venezuelano, che da sempre condivide i valori occidentali. A questo punto pare evidente come i cittadini venezuelani, la cui libertà decisionale è stata limitata già per troppo tempo, vadano accompagnati e assistiti per invertire il flusso di questo regime autoritario e antidemocratico, che ha danneggiato il Paese sotto tutti i punti di vista. È necessario coinvolgere la comunità internazionale, tramite le sue istituzioni, nell'assicurare la partecipazione alle elezioni del 2024 anche ad attori politici esterni al regime di Maduro, rilasciando i prigionieri politici, al fine di permettere lo svolgimento di una competizione elettorale libera, equa e inclusiva. Mi lasci, Presidente, ringraziare per suo tramite il presidente della Commissione affari esteri e difesa, senatrice Stefania Craxi, e tutti i membri della Commissione che unitamente hanno lavorato su questa risoluzione, per essere di supporto alle prossime elezioni, che tutti auspichiamo possano essere democratiche per il Venezuela, per i venezuelani e per i 160.000 italiani che abitano in quel meraviglioso Paese. Annuncio quindi il voto favorevole del Gruppo Lega su questa risoluzione.

il Gruppo parlamentare Partito Democratico voterà a favore di questa risoluzione e lo farà - mi sembra di capire, a sentire le dichiarazioni precedenti - in buona compagnia,

ma soprattutto ci ringraziamo a vicenda, perché è importante che, sulle grandi questioni di politica internazionale, ci sia la capacità di realizzare l'unità del Paese.

dopo una prima fase di contrapposizione a 360 gradi, gli Accordi di Barbados, stipulati il 17 ottobre 2023, hanno suscitato in tutti noi la speranza che finalmente si andasse verso un corso democratico. Quegli accordi erano il frutto di trattative segrete, in parte mediate anche da Paesi esteri, tra la maggioranza e l'opposizione. L'opposizione, nei mesi successivi, dopo lunghi periodi di divisioni - qui noi guardiamo alle responsabilità del regime, che sono enormi, ma l'opposizione per lungo tempo ha marciato completamente divisa - ha realizzato una straordinaria unità attorno a una donna, Maria Corina Machado, che quando io incontrai a più riprese alla fine del 2019 e precedentemente nel 2016, quando andai in Venezuela, rappresentava una piccola parte dell'opposizione. Tenendo duro contro tutto e contro tutti, María Corina Machado ha realizzato l'unità dell'opposizione. L'abbiamo ascoltata in Commissione affari esteri, naturalmente via telefonica. Il risultato di tutto questo è stato, dopo gli accordi di Barbados, la possibilità di elezioni presidenziali, quelle di cui stiamo discutendo.

almeno due candidati, e i candidati dell'opposizione in un Paese parademocratico li sceglie il Presidente in carica, ma l'opposizione. *(Applausi)*. Infatti l'opposizione è andata a votare in primarie che hanno avuto un'affluenza straordinaria scegliendo Maria Corina Machado.

ai milioni di origine italiana che vivono in Venezuela, ma anche alla povera gente, ai cattolici venezuelani, agli uomini, alle donne e ai giovani di quel Paese, molti dei quali sono costretti ad espatriare nei Paesi vicini - è che si è persa un'occasione straordinaria per restituire al mondo il Venezuela. Ricordate, colleghi: all'inizio degli anni Sessanta il Venezuela era meta della nostra emigrazione, perché era uno dei Paesi emergenti del mondo sotto il profilo economico e imprenditoriale, con risorse straordinarie. Tutto questo se ne è andato. Credo Credo che non serva a molto rivolgere appelli a Maduro, perché quello che sta capitando è la dimostrazione della negazione di princìpi basilari su cui si regge il processo democratico. Ho incontrato il Presidente venezuelano

Presidenti che Maduro ha salutato come discontinuità rispetto ai precedenti Presidenti, e sono tutti appartenenti alla sinistra. parliamo di sinistra non europea, ma di sinistra-sinistra, quella sudamericana, una cosa che ha anche una discontinuità rispetto al tema del socialismo europeo. tutti quei Paesi hanno condannato fermamente quello che sta capitando. Dunque, il problema forse non è l'Italia, non è l'Europa, non sono gli americani: il problema è il mondo, che vede con preoccupazione questo ulteriore atto di prevaricazione. I candidati non vengono scelti da chi vuole fare elezioni di comodo; sono gli elettori che si scelgono i candidati. Se poi Corina Machado vince o perde, è una cosa che fa parte del processo democratico, ma non può essere una cosa che viene decisa a tavolino. Qui si sono esclusi i candidati che potevano vincere,

la quale ha fatto un passo indietro, con grande disponibilità, forse superiore a quella che avremmo avuto noi. si è messa a lato e c'è stata la designazione di una nuova candidata, sempre un'altra donna, una professoressa molto credibile. Che cosa è successo?

Colleghi, è giusto votare questa risoluzione. È una pagina triste e noi non abbiamo alcuna soddisfazione nel procedere a quest'atto. Noi vorremmo che il Venezuela, grande Paese, con un popolo meraviglioso, venisse restituito alla comunità internazionale e riprendesse quel ruolo che tradizionalmente ha avuto. Voglio fare un'ultima considerazione, un'ultima considerazione, rivolta a Chavez e al *chavismo*. Francamente, con tutta la generosità possibile, io non posso certo essere considerato un fan del *chavismo*. Chavez, ha vinto il processo democratico, perché aveva una convinta e reale adesione del popolo venezuelano. I processi elettorali di Chavez sono stati veri processi elettorali. La sua politica può essere stata anche pessima,

è finita anche quella fase lì; una fase in cui, nella contrapposizione durissima, il potere, però, era legittimato dalla gente. Oggi, in termini di legittimazione, non c'è più nulla. Il Venezuela rischia di essere

Signor Presidente, onorevoli senatori, dopo undici anni di Governo Maduro il Venezuela andrà al voto, il prossimo 28 luglio, con il concreto sospetto, anzi con la certezza, che queste elezioni prendano di nuovo una deriva contraria alla democrazia, considerando innanzitutto il fatto che alla principale candidata delle opposizioni e vincitrice delle primarie di ottobre, Maria Corina Machado, è stato impedito di partecipare alla competizione. La *dama de acero* è stata praticamente eliminata dalle elezioni, con il divieto di candidarsi a cariche pubbliche, tramite una sentenza di esclusione emessa da una Corte suprema di giustizia priva di giurisdizione penale. La sentenza è il risultato di un processo oscuro, senza l'esercizio del diritto alla difesa, ed è costellata di vizi procedurali. Oltre a Maria Machado, il regime ha interdetto dalla competizione politica altre personalità di spicco dell'opposizione, come Capriles e Superlano. Altri, come Camacaro, Freites, Lopez e Venegas sono stati catturati e fatti sparire dalle forze repressive della dittatura. Gli altri attivisti vengono perseguitati, anche con false accuse e mandati di arresto. Numerosi Paesi sudamericani hanno espresso preoccupazione per i risultati delle prossime elezioni, soprattutto dopo l'esclusione delle opposizioni. Anche noi siamo fortemente preoccupati che in questa tornata non vengano garantiti il pluralismo e lo Stato di diritto. Perciò, vogliamo ribadire ancora una volta che per quest'Aula il diritto alla partecipazione in politica è sacrosanto ed è il punto cardine di ogni civiltà. All'opposizione, a tutte le opposizioni, devono essere riconosciuti i diritti civili e il necessario spazio democratico. Il Senato italiano, perciò, non poteva non esprimersi, perché le elezioni del Venezuela si presentano come un bivio cruciale per il futuro del Paese sudamericano, ma anche per gli interi equilibri geopolitici mondiali. Se il Venezuela sarà in grado di intraprendere la strada di elezioni libere e nel pieno rispetto del pluralismo, potrà andare finalmente nella direzione di un domani economicamente più prosperoso, socialmente avanzato e certamente più pacifico per il Paese e per il mondo. Se l'opposizione riuscirà a emergere vittoriosa, per il Venezuela potrebbe finalmente prospettarsi un cambiamento a livello sociale, politico ed economico. Maduro è in carica dal 2013, nonostante l'ultima volta sia andato a votare solo il 30 per cento dei cittadini e nonostante oggi, secondo i sondaggi, la sua popolarità non superi il 15 per cento. Durante gli undici anni del suo Governo, il Venezuela ha vissuto un'inflazione del 286 per cento; un quinto della popolazione (quindi 6 milioni di persone) ha lasciato il Paese. L'era Maduro è perciò quanto di più distante dall'essere un'epoca d'oro, guidata da un supereroe che tutela il popolo. I venezuelani non hanno visto nessun factor "M", come piace chiamarlo (a Maduro ovviamente), che li abbia realmente sollevati dall'attuale disastro economico, di proporzioni tali da far rientrare il Venezuela per due anni consecutivi tra i dati più alti del *misery index*. index*. Ci chiediamo allora con che coraggio Maduro oggi lanci la sua campagna elettorale, pubblicando la serie animata del «Super Bigote», un Clark Kent col baffo che lotta contro gli oppositori politici e il terribile impero americano. Ma quale Superman! Forse più un Super Mario Bros, che ogni volta che fa scomparire un avversario con un calcio crede di racimolare una sparuta moneta di consenso e invece contribuisce ad aggravare la crisi sociale e umanitaria in corso. Da che cosa dovrebbe difendere i venezuelani, se non da se stesso, dal suo regime, dalla sua oligarchia di chiaro stampo socialista, che sta piegando con la violenza e con la fame un intero popolo e che ha ceduto alle sirene di Russia e Cina, che già vennero in soccorso di Maduro nel 2019, ponendo il veto al Consiglio di sicurezza dell'ONU alla mozione americana che chiedeva elezioni libere e finalmente credibili? Insomma, nonostante il 60 per cento dei venezuelani auspichi l'immediata destituzione di Maduro, a riconoscere oggi un Presidente rimasto al potere grazie ai voti di scambio, ai brogli, all'astensione da *record*, alla corruzione dell'esercito, alla gestione di traffici illeciti e a una popolazione stremata stremata dalla crisi e quindi incapace di ribellarsi, a sostenere un Presidente perciò chiaramente frutto di elezioni fraudolente ci sono - pensate un po' - Cina, Russia, Cuba, Nicaragua, Bolivia e Turchia, ovvero dittature già riconosciute come tali. Non solo: anche Hamas ed Hezbollah hanno preso una chiara posizione, dichiarando il proprio sostegno al *leader* del PSUV, perché nutrono legami di stretta collaborazione con i cartelli della droga e degli apparati paramilitari. A ciò si aggiunga che in questo momento Maduro è sotto inchiesta della Corte penale internazionale per crimini contro l'umanità, perché sono documentate almeno 1.521 vittime di tortura e 7.500 vittime di trattamenti crudeli, inumani e degradanti, tra cui anche centinaia di bambini. Le forze di sicurezza e i gruppi armati filogovernativi, i *colectivos* (un nome così amato anche da taluni in Italia), hanno ripetutamente attaccato le manifestazioni del 2014 con *raid* violenti, pestaggi e sparatorie a distanza ravvicinata. Gli agenti della Faes e di altre unità militari e di polizia hanno ucciso e torturato impunemente nelle aree più povere. Tutte cose che già vediamo esattamente in dittature decennali come, appunto, Cuba e Iran. Nessuna Nessuna posizione neutrale è accettabile. Nessun partito può incorrere nel grave errore di definirsi amico di un regime sanguinario, come credo qualcuno tra questi scranni ha fatto in passato, scrivendo una pagina triste e opaca della nostra storia. Di fronte a quella che di fatto si rivela pienamente come una dittatura vile e assassina, la voce di Fratelli d'Italia, di questo Governo, di quest'Assemblea e, più in generale, quella di tutti gli uomini liberi, che credono nella democrazia e nella dignità della persona, non può che schierarsi da un'unica parte: quella del popolo e quella della libertà. Concludo, Presidente, salutando con un abbraccio pieno di speranza innanzitutto Maria Claudia Lopez, rappresentante di Maria Corina Machado, le associazioni degli esuli venezuelani in Italia e, tra questi, quella presente oggi in Senato, «Casa Italo-Venezuela» e poi, ancora, «Venezuela: la piccola Venezia», «Unione Italo-Venezuelana» e «Venezuela in Toscana». infine il voto favorevole di Fratelli d'Italia, con un unico grande auspicio: *Venezuela libre ahora*.

colleghi, prima di rispondere in merito ad alcune critiche avanzate dai colleghi dell'opposizione, desidero ringraziare il presidente della 7ª Commissione, senatore Marti, e tutti i componenti per il lavoro svolto. Sulle critiche avanzate e soprattutto sul contenuto della riforma preciso che il nostro intervento è volto a sostituire, per la valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni nella scuola primaria, dei giudizi finalmente chiari e comprensibili che non sopprimono la descrizione del percorso umano e pedagogico delle alunne e degli alunni (aspetto per noi fondamentale e imprescindibile). Infatti, i giudizi sintetici devono essere correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento, che costituisce la griglia alla quale, con modalità più comprensibili per le famiglie, si dovrà continuare a fare riferimento. Inoltre, Presidente, desidero ricordare, tramite la sua persona, alla senatrice Malpezzi che siamo intervenuti su uno dei decreti legislativi della cosiddetta

che ha introdotto nel primo ciclo di istruzione (e quindi anche nella scuola primaria) non il giudizio sintetico, sentite bene - addirittura una valutazione espressa con un voto in decimi. Quindi capisco, signor Presidente, che spesso la memoria ci inganna. Inoltre, voglio rispondere ai colleghi dell'opposizione che hanno avanzato in Commissione critiche sotto il profilo del metodo. Faccio presente che questa maggioranza è intervenuta, a differenza del passato, nel modo più lineare possibile. Stiamo esaminando un disegno di legge che, dopo un percorso di consultazione e di dibattito anche politico svolto dal ministro Valditara e dal suo Ministero prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, sta seguendo, senza nessuna scorciatoia procedurale, un *iter* ordinario. Quindi non corrisponde a verità dire che le disposizioni introdotte da questo disegno di legge intervengono direttamente sullo Statuto delle studentesse e degli studenti. Questo disegno di legge, come è giusto che sia, introduce nuovi principi e criteri per l'adeguamento del predetto Statuto, che è contenuto in un regolamento che sarà modificato nel rispetto, ribadisco, di tutte le procedure, oltre che svolgendo tutte le consultazioni che sono previste dalla legge. Sorprende anche, signor Presidente, che queste critiche vengano proprio da chi era al Governo e ha modificato, con un vero colpo di mano parlamentare, quindi con un emendamento inserito in una legge di conversione di un decreto-legge, la disciplina della valutazione degli studenti, che noi invece stiamo provando a riscrivere alla luce del sole ed in esito ad un pubblico confronto parlamentare. Mi riferisco in particolare a quando, con il ministro Azzolina, si intervenne con un emendamento al decreto-legge n. 22 del 2020 per introdurre il giudizio descrittivo in luogo di quello in decimi - si badi bene: in decimi - voluto dal ministro Fedeli. E allora dico: PD e MoVimento 5 Stelle, che si sono divisi al tempo rispetto alle loro opinioni, oggi sono invece allineati. Evviva la loro coerenza. Si è parlato di differenza tra autorità ed autorevolezza. Signor Presidente, conosciamo benissimo la distinzione ed è proprio su questo che si basa questo disegno di legge disegno di legge che vuole sostituire la fallimentare sospensione *tout-court*, intesa come semplice allontanamento dalla scuola, un atto demotivante, un residuato di un potere autoritario che non si vuole più. Infatti siamo intervenuti in modo più fattivo, con più scuola, attraverso attività scolastiche di riflessione e di apprendimento, su temi legati ai comportamenti che hanno causato quel provvedimento, per raggiungere il vero obiettivo, che per noi è importantissimo, che è la vera e fattiva maturazione e responsabilizzazione dell'alunno. Altra critica avanzata dal collega senatore Verducci, è che per questa maggioranza ogni contestazione è un reato. E allora, signor Presidente, tramite la sua persona rispondo al collega: noi non puniamo chi contesta, ma chi devasta la scuola. L'obiettivo di questo disegno di legge è proprio quello di ripristinare la cultura del rispetto, di contribuire ad affermare l'autorevolezza dei docenti e di riportare serenità nelle nostre scuole. Ecco perché si è intervenuti sui criteri di valutazione del comportamento nelle scuole secondarie. non c'è nulla di arbitrario, non c'è nulla di punitivo in questo disegno di legge. C'è semplicemente l'obiettivo di tutelare e dare autorevolezza e decoro a questa grande istituzione. Infine, Presidente, si è criticato questo Governo perché nulla ha fatto sulla povertà educativa, sulla dispersione scolastica che non si capisce e non si conosce i concetti di una scuola aperta ed inclusiva. Chiudo con un piccolissimo riassunto, ricordando l'investimento 1.4, «Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali

decreto Agenda Sud, il decreto-legge Caivano sulla dispersione scolastica, per chiudere con il Piano estate 2024. Signor Presidente, capisco che le opposizioni fanno finta di dimenticare, visto che investimenti così importanti nei precedenti Governi erano solo un sogno, oppure - peggio - venivano destinati ad obiettivi ancor più scellerati, inefficaci e fallimentari.

chiedo di illustrare tutti gli emendamenti presentati dal nostro Gruppo all'articolo 1 del disegno di legge in discussione, come consentito dal nostro Regolamento. Onorevoli colleghe e colleghi, stiamo discutendo un disegno di legge che riteniamo essere pieno di criticità; scusate la mia durezza, ma non servono troppi giri di parole. Con queste norme che oggi ci presentate, la scuola italiana rischia di fare un passo indietro di decenni e di smantellare quanto è stato fatto sino ad oggi per l'istruzione e il rafforzamento di tutta la comunità educante. Lo sforzo del nostro Gruppo per costruire una linea emendativa è dipeso proprio da questo: avremmo voluto cancellare e riscrivere le norme che partono da assunti sbagliati per arrivare a esiti non condivisibili. Con gli emendamenti che oggi saranno messi in votazione cerchiamo quindi di porre rimedio alle molte storture presenti nel testo, a partire da una domanda: una dimensione così complessa e astratta come la vita a scuola delle studentesse e degli studenti può essere davvero ridotta ad un voto, ad un numero? il modello di una scuola come luogo di formazione della cittadinanza, di dialogo e condivisione può essere smantellato, come sembra voler fare il Governo, per far posto sempre ad un modello punitivo? Purtroppo questi dubbi sono diventati certezze anche durante i lavori in Commissione. Non contenti di rivedere il sistema di valutazione del comportamento degli studenti nelle scuole medie e superiori, si è anche inserito, con un subemendamento del Governo, un sistema di valutazione degli alunni alle scuole elementari che ci fa tornare indietro di dieci anni, se non di più, al sistema numerico. Diciamolo con chiarezza: la volontà di cancellare il voto descrittivo nelle scuole di primo grado fa parte dello stesso disegno punitivo che pervade tutto questo provvedimento; esattamente il contrario di quanto espresso anche durante le audizioni dai tanti soggetti del mondo della scuola, che chiedevano, all'opposto, di rafforzare i percorsi di confronto e condivisione. Con i nostri emendamenti chiediamo di non ritornare al voto numerico, seguendo un principio chiaro: la scuola non serve a selezionare i migliori, semmai a non lasciare indietro nessun ragazzo nel percorso di crescita. Nella costruzione degli emendamenti all'articolo 1 siamo partiti dall'assunto che garantire autorevolezza agli insegnanti nella loro funzione pubblica e accrescere il riconoscimento sociale del loro ruolo, che riteniamo essere un dovere dello Stato, non significa rafforzare il loro potere giudicante verso gli studenti, semmai il contrario. Dovremmo investire sulla valorizzazione della loro professione, sul superamento del precariato. Vengo quindi ad una questione ancora più importante e più distorsiva contenuta in questo disegno di legge: il voto numerico in condotta. Noi diciamo una cosa semplice: il voto in condotta in decimi è già stato utilizzato diverse volte nella storia e non ha restituito grandi risultati; inoltre, in quanto numero, fotografa una situazione e non opera un'azione di cambiamento. La scuola deve invece assumere il compito di liberare gli studenti da condizionamenti negativi; ancora peggio, poi, quanto previsto nelle scuole superiori, con la scelta di assegnare a uno studente il numero massimo di crediti all'esame di Stato solo perché ha nove in condotta: è un errore, perché è uno sbilanciamento del valore del voto in condotta rispetto al resto del profitto degli studenti e delle studentesse. Vado avanti, signor Presidente, segnalando che questa maggioranza, con il disegno di legge in esame, sembra aver dimenticato ancora oggi che la scuola è retta dal principio dell'autonomia. Le norme di questo disegno di legge - e penso all'obbligo di bocciatura senza il 6 in condotta - in alcuni casi sono troppo coercitive, togliendo ai consigli di classe la facoltà di affrontare le valutazioni caso per caso, individualità per individualità. Con le nostre proposte chiediamo di ridare ai consigli di classe il loro ruolo, perché conoscono i ragazzi e le ragazze ed è importante che abbiano modo di apprezzarne e riconoscerne i miglioramenti anche nel profitto e nella valutazione, eventualmente Sulla condotta però il Governo fa ancora peggio, perché costruisce un castello di norme stringente, tutto orientato a trasformare la scuola in un luogo di punizione, senza tener conto della comunità educante, che ruota attorno alle studentesse e agli studenti.

noi proponiamo il coinvolgimento delle famiglie dei ragazzi e delle ragazze con rendimento in condotta scarso e dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse, prima di arrivare ai provvedimenti disciplinari. Peggio: viene modificato lo Statuto scolastico senza ascoltare le organizzazioni studentesche; addirittura, si è arrivati a pensare a provvedimenti disciplinari che schiacciano l'orientamento della valutazione tutto sull'aspetto coercitivo. Si pensi all'idea di rimandare a settembre i ragazzi con 6 in condotta e soprattutto ai progetti di cittadinanza solidale, che spingono la punizione anche fuori dai confini dell'istituto scolastico. Signor Presidente, chiediamo di modificarli, perché assomigliano alle pene inflitte per i reati minorili. Riteniamo inoltre sbagliato sospendere il giudizio degli studenti con 6 in condotta e rimandarli a settembre: su questo proponiamo che, al fine di stimolare le studentesse e gli studenti alla partecipazione attiva e al senso di responsabilità nei confronti della comunità scolastica, intesa come comunità educante, il Ministro dell'istruzione e del merito adotti linee guida per l'insegnamento di cittadinanza e Costituzione, previa consultazione del Forum delle associazioni studentesche e delle rappresentanze degli studenti. Esiste quindi un'altra strada per il presente e il futuro delle nostre scuole? Sì: abbiamo cercato di tracciarla, proponendo di mettere da parte questo sistema di norme e di punizioni per recuperare invece la dimensione sociale, educativa e inclusiva della scuola. Soprattutto, proponiamo di modificare questo provvedimento per cercare di costruire una legge che sia davvero utile ai nostri studenti e alle nostre studentesse. Lo abbiamo visto in questi mesi con i movimenti studenteschi e la campagna migliaia di ragazze e ragazzi in tutta Italia si sono mobilitati per chiedere risorse e attenzione sul tema della salute mentale. Come Partito Democratico, abbiamo chiesto che le scuole si aprano ai percorsi per il benessere psicologico degli studenti e degli insegnanti. Chiediamo anche di avviare un progetto sperimentale in tutti gli istituti con lo sportello psicologico, oggi presente già in alcune scuole, con risultati molto positivi. positivi. Con i nostri emendamenti, proponiamo il modello di una scuola che non si ispiri al paradigma della punizione, ma recuperi invece i valori dei grandi educatori del nostro Paese. Per questo motivo, condividiamo le modifiche sulle sezioni a metodo didattico differenziato Montessori, ma riteniamo sia davvero poco per rendere accettabile il testo di legge che ci viene proposto. Occuparsi del benessere psicologico dei nostri giovani pensare la scuola come luogo di formazione dei cittadini di domani è la priorità per il Partito Democratico. Abbiamo cercato di rafforzare questo impegno anche prevedendo con un altro emendamento un sostegno all'intera comunità scolastica, con la figura di un sociologo negli istituti, capace di porre un freno alla povertà culturale ed educativa che attraversa molti territori del nostro Paese. Non si risolve il disagio giovanile con l'ossessione per la condotta; semmai si ottengono gli effetti contrari. Siamo preoccupati per il clima che si respira nel Paese; abbiamo assistito ad episodi nelle scuole italiane che sembrano anticipare lo stesso atteggiamento repressivo che ritroviamo nelle norme di questo disegno di legge. A Modena, la mia città - lo ricordava ieri il senatore Verducci - uno studente è stato sospeso per dodici giorni solo per aver fatto un'intervista in cui segnalava le criticità dell'istituto scolastico. Ho presentato un'interrogazione al ministro Valditara, generalmente fin troppo loquace; ma, davanti a questi fatti, non ha ancora deciso di rispondere. Signor Presidente, arrivo alle conclusioni della mia illustrazione. Gli emendamenti del Partito Democratico provano a disegnare i tratti di una scuola che sia sempre più ancorata ai principi del dialogo e della condivisione. Siamo convinti che dobbiamo tutti lavorare perché la scuola diventi sempre più un luogo dove gli studenti e le studentesse vanno volentieri, in cui possono costruire percorsi di cittadinanza solidale e di inclusione sociale. Una scuola dove ogni studentessa e studente possano imparare a conoscere il proprio paesaggio emotivo, possano imparare a conoscere e ad argomentare la complessità di una comunità. La scuola come luogo e tempo dove possono trovare risposte le tante domande che ogni studente e studentessa si pongono per capire il mondo nel quale andranno ad abitare e a vivere.

tutta la parte descrittiva con gli indicatori. In quella discussione, che molti di noi in quest'Aula avevano comunque condiviso, si raccontava della necessità di superare la valutazione precedente, fatta solo di lettere, per arrivare tramite a quella che doveva essere una vera e propria valutazione formativa, che è stata poi in effetti realizzata. Ciò perché crediamo nel coinvolgimento di tutto il consiglio di classe, perché riteniamo che la valutazione sia una scelta del consiglio di classe, che deve tener conto che deve tener conto di tutti i fattori che riguardano la crescita della studentessa e dello studente, le difficoltà, gli *step*, i passaggi, le conquiste effettuate, tutte le paure superate: questo è educare. È per tale motivo che, ancora una volta, l'emendamento in esame mette in evidenza questi elementi, rispetto ai quali noi continuiamo a ribadire che rafforzano la cittadinanza e la partecipazione delle bambine e dei bambini del nostro Paese, semplicemente perché in questo modo riescono a crescere meglio.

Signora Presidente, io posso capire - e interverrò successivamente sull'emendamento aggiuntivo che ci apprestiamo a votare dopo questo ordine del giorno un parere negativo. Ormai siamo abituati al fatto che non siete capaci di valutare nel merito nessuna questione e che, aprioristicamente, sapete dare solo pareri negativi. Ma persino su un ordine del giorno mi sembra veramente

Dell'idea di offrire un supporto agli studenti, uno spazio di dialogo, un luogo dove possano aprirsi se n'è parlato già diverse volte e, seppure in termini diversi, i pareri erano stati diversi. Questo ci fa pensare che neanche leggiate gli ordini del giorno e gli emendamenti proposti dall'opposizione e i vostri pareri siano aprioristici. Questa è una vergogna, e non per la dignità del lavoro dei parlamentari, ma per i cittadini italiani, per le persone che si aspettano che siate in grado di governarlo, questo Paese, e non solo di prendere delle decisioni ottuse e sulla base di giudizi aprioristici. *(Applausi)*. Non è questo quello che meritano i nostri studenti, non un atteggiamento repressivo e non capace di capire le difficoltà in cui versano. Non potete valutare tutto con il metro del giudizio della repressione della punizione. Invece è solo questo quello che mettete in campo per i nostri giovani. In realtà, è l'unica cosa che siete capaci di mettere in campo in qualsiasi settore. Ma, quando questo avviene nei confronti di di quello che sarà il futuro del Paese, ha un peso ancora peggiore. Non siete in grado di valutare la scuola come comunità educante, che è quello che deve essere. Siete capaci solo di oppressione, ed è un male. Mi domando che razza di infanzia avete avuto, se l'unica cosa che conoscete è questa.

Colleghi, per cortesia. PIRRO *(M5S)*. Penso che siamo tutti consapevoli delle difficoltà che affrontano ogni giorno i nostri giovani. Penso che tutti dovremmo ricordarci quello che in quest'Aula, nella scorsa legislatura, ci siamo detti a valle del *lockdown* e della pandemia a proposito dei nostri ragazzi e di come possa essere stato traumatico per loro affrontare quei difficili momenti. Ricordo che è stato traumatico anche per gli adulti, in quanto credo nessuno di noi abbia ricordo ricordo di eventi simili accaduti nella propria infanzia, nell'adolescenza. Quindi, se per noi il *lockdown* e la pandemia sono stati un trauma, a maggior ragione lo sono stati per i nostri giovani che non avevano gli strumenti...*(Brusìo).* Presidente, gradirei non avere brusìo nelle orecchie, se è possibile. Ci siamo detti che, forse, dopo la pandemia saremmo stati tutti migliori, ma pare che ciò purtroppo non sia Di sicuro è avvenuto qualcosa nel nostro Paese, perché ci siamo resi conto dell'importanza di un supporto psicologico e della necessità di aiutare prevalentemente i nostri ragazzi, ma forse ciò servirebbe anche agli adulti. adulti. La nostra Costituzione ci ricorda il valore educativo delle istituzioni scolastiche e l'importanza di un atteggiamento solidaristico nei confronti dei più fragili, anche se dai provvedimenti che emaniamo sembrerebbe che non tutti abbiamo ben presente questo concetto. Ho partecipato ieri alla Camera dei deputati a una conferenza stampa sui risultati di uno studio sui

Tutti ci siamo detti che non bisogna intervenire sempre con *bonus,* che bisogna fare interventi strutturali, che dobbiamo aiutare i nostri giovani e che spesso gli atteggiamenti aggressivi possono essere prevenuti. Prevenzione: questa parola tanto manca nel nostro Paese e nei nostri atti parlamentari, e mi riferisco a quelli che vengono approvati, perché in quelli proposti dalle opposizioni è ricorrente, ma sottovalutata. Per queste ragioni, l'emendamento proponeva un intervento strutturale nelle nostre scuole, con uno sportello di *counseling* e supporto ai nostri giovani, per evitare di doverli poi punire a valle. Le punizioni arrivano sempre dove si è fallito nell'intervento educativo, ma si stenta a farlo stenta a farlo capire. *(Applausi)*. Per queste ragioni, continuiamo a proporre in quest'Aula - e continueremo finché non diverrà legge dello Stato, magari con una diversa maggioranza - la proposta di istituire in tutte le scuole di ogni ordine e grado uno sportello di supporto psicologico, *counseling* e ascolto per i nostri giovani che ne hanno bisogno. questa maggioranza e questo Governo sono completamente sordi al grido di aiuto che arriva dai giovani.

Presidente, colleghe e colleghi, membri del Governo, non entro nei particolari del provvedimento, se non

Quello che mi preme dire stamattina come neuropsichiatria e anche come padre e nonno

un discorso serio, se vogliamo intelligente, di contrapposizione in ambienti dove l'apprendimento, la serenità, la condivisione, l'inclusione vivono. Non esiste la cultura dei professori e dei maestri contro i ragazzi, i bambini e le bambine e viceversa. Questa visione "paleo" di sinistra fa male a tutti, intanto perché è irreale e poi perché, casomai, il nostro ruolo è quello di ridurre al minimo le conflittualità. Nell'apprendimento due sono le cose che contano: la dolcezza di chi ha la possibilità di trasferire competenze e la fiducia di chi le riceve. Un buon padre e una buona madre non possono non essere autorevoli e rispettati, certamente rispettosi dei figli, perché altrimenti si creano una rabbia e una sfiducia che non fanno bene a nessuno.

giovanile di grande sconquasso, di grande perdita di certezze e di messaggi contrastanti, qualche volta manifestano impropriamente il loro disagio, diventando persino violenti sugli insegnanti. Questa realtà non ci deve far dire: siamo con questi o siamo con quelli. Non dobbiamo esercitare il tifo per qualcuno contro qualcun altro. Non c'è l'uno contro l'altro, ma esiste un sistema fatto di adulti, bambine, bambini e ragazzi che vogliono il massimo della serenità, altrimenti non si cresce mentalmente. Ve lo garantisco, occupandomi da mezzo secolo e oltre di apprendimento e salute mentale: chi è più fragile, chi deve apprendere deve avere fiducia e rispetto, non deve avere un contropotere, perché gli sconquassa il cervello. Quando ascolto alcuni interventi dell'opposizione, come l'ultimo, mi riempio di amarezza, di sconforto,

sentisse un senatore della Repubblica offendere reiteratamente chi non la pensa allo stesso modo, quale apprendimento avrebbe, che fiducia avrebbe nelle istituzioni, in questa pornografia della politica? Allora, Presidente, con tono sommesso dico che, votando favorevolissimamente questo provvedimento, non posso non esprimere preoccupazione di questo atteggiamento schizofrenico, nel quale si tende a fare una politica buona e buonista, dicendo cose oscene e crudeli. Vede, Presidente, diceva qualcuno molto più bravo di me che l'inferno è lastricato di buone intenzioni. Io dico che stamattina in quest'Aula qualcuno che dice di avere buone intenzioni in realtà guarda con affetto l'inferno. Noi non vogliamo questo, ma vogliamo che i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze vivano l'insegnante e le famiglie come se fossero una squadra, non in competizione, ma per apprendere tutti - anche gli insegnanti - il valore della diversità delle idee, il valore di competere per migliorare le proprie *performance.*

sicurezza e non buonismo d'accatto che non serve a nessuno. Io odio la contrapposizione generazionale artatamente creata: non ci sono buoni e cattivi, esistono soltanto persone di età diverse, con i loro dolori, con le loro gioie, con le loro frustrazioni e le loro conquiste. È un momento difficilissimo. Si parla troppo di morti di guerre e meno di pace e voglia di vivere, ma è nostro compito migliorare per quanto possiamo il sistema, portando serenità anche in quest'Aula e non delegittimazione

la prima considerazione che voglio fare oggi in quest'Aula è quella che, sulla scia degli episodi violenti e delle aggressioni che ci sono stati in alcune scuole, questo Governo legifera sull'onda emotiva ed emergenziale. Continuate così, che andiamo a sbattere completamente! *(Applausi)*. Non c'è una risorsa in più sulla scuola, sul diritto allo studio

positivi e soprattutto guardando alla fotografia impietosa che ci viene dall'Istat. I dati dell'Istat ci dicono che, dopo il Covid, questa generazione e soprattutto le politiche di *welfare* sono entrate in una fase di collasso totale, perché non c'è stato alcun investimento sul disagio giovanile

che il Governo dovrebbe farsi è come agire sulle politiche di prevenzione, non con politiche che vanno sempre in un'unica direzione, quella di essere punitive e repressive. Come si fa a legiferare sempre in questo modo? È il motivo per cui noi di Italia Viva abbiamo cercato di spiegare in tutti i modi che bisogna andare in un'altra direzione, quella degli investimenti. Quando parliamo di scuola - e mi dispiace, ma questa è la realtà siamo fermi agli ultimi investimenti sul sistema scolastico dei tempi del Governo Renzi, con la cosiddetta legge buona scuola. Siamo fermi ancora lì. lì. Perché ogni volta dovete sempre demolire tutto e ricominciare daccapo, invece di partire dalle buone pratiche adottate dai Governi precedenti, che stavano portando buoni risultati? *(Applausi)*. Dopodiché, si può sempre migliorare, ma non cancellare tutto. Scusate,

Italia Viva-Il Centro-Renew Europe ha parlato sempre in quest'Aula di costruire invece un nuovo patto educativo tra famiglie e scuola. Non possiamo pensare di delegare tutti i problemi alla scuola, ma non possiamo neanche lasciare le famiglie da sole, che spesso sono monogenitoriali, e hanno bisogno di aiuto e sostegno. Ecco perché una politica attenta ai bisogni della cittadinanza, una politica attenta a difendere un diritto sancito dalla Costituzione, come il diritto allo studio.

una programmazione, dove si continua invece ad aumentare le tasse e a non investire nei pilastri che riguardano i sistemi di politica sociale e di *welfare* sui territori. E ora sui territori. E ora le Regioni, indipendentemente dal colore politico, e gli enti locali vi stanno lanciando un grido d'allarme in maniera molto chiara, perché non si stanno facendo investimenti in quella direzione. E il sistema inevitabilmente collassa. collassa. Siccome noi non siamo mai ideologici e populisti, ma siamo riformisti fino in fondo, siamo sempre pronti a collaborare con il Governo e con il Parlamento, quando ci sono provvedimenti attenti alle politiche sociali. Ma in questo caso

all'interno di questo provvedimento, fossero prese delle precauzioni rispetto all'utilizzo, a volte sproporzionato, dei cellulari in aula. *(Applausi)*. Questo poteva essere un investimento importante, in un nuovo patto di collaborazione, di dialogo e di confronto tra la scuola, la famiglia, i genitori e gli studenti (tutto quello che ovviamente non prevede come strumenti didattici). Se vogliamo parlare seriamente di questo tema e non fare il solito provvedimento sull'onda emotiva o emergenziale, parliamo di come

extrascolastiche, ad esempio utilizzando lo strumento, a noi molto caro come partito, di aumentare l'attività motoria nelle scuole, che abbiamo visto funzionare benissimo come contrasto a tutti i tipi di dipendenza e per creare inclusione sociale. Questa è la scuola. La scuola è quella che non vuole lasciare indietro nessuno, che fa politiche coraggiose di educazione di attenzione ai territori. Le diseguaglianze sociali, economiche e culturali sono aumentate ancora di più dopo il Covid, e lo sappiamo benissimo. Gli investimenti li dobbiamo fare su questo: come ridurre le distanze e le diseguaglianze. Parliamo di come contrastare, per esempio, la dispersione scolastica - noi vorremmo parlare di questi temi - di come contrastare il continuo aumento della povertà educativa e anche digitale in molte famiglie. Queste sono le cose di cui avremmo voluto parlare oggi con questo provvedimento. Il 60 per cento delle scuole italiane non ha una palestra. Ma vi rendete conto? Stiamo parlando di DEF, di PNRR e non parliamo di questo, di edifici scolastici fatiscenti, di strumenti didattici e informatici che non sono all'avanguardia, di pochi laboratori in molte scuole. Parliamo di questo, di come investiamo nella scuola, di come investiamo nella sanità, di come aumentiamo, per esempio, lo sportello di ascolto dello psicologo a scuola. Abbiamo presentato anche una proposta di legge, che mettiamo a disposizione di tutto il Parlamento, con cui si prevede la reintroduzione del medico scolastico come altro presidio di prevenzione, per capire quali sono le paure, le insicurezze e i disagi che oggi hanno i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Per tutti questi motivi, siamo costretti oggi - lo dico con rammarico - ad esprimere un voto contrario, proprio perché si è scelta la strada punitiva e repressiva, invece di andare incontro ai problemi reali della scuola *(Applausi)*, ad una valutazione attenta che deve prevedere un giudizio complessivo. Ad ogni ragazzo e ragazza bisogna dare una possibilità, perché in ognuno di loro ci sono delle opportunità straordinarie e dei talenti nascosti. Non può essere il voto di condotta, che considero

e dell'Istituto di istruzione superiore «Olivelli Putelli» di Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia.

attorno al quale in piena pandemia si discusse molto. Erano - lo ricordiamo tutti - i giorni più difficili per la scuola italiana, obbligata a scelte mai nemmeno immaginate fino a quel momento. Avevamo la percezione forte che quella situazione inedita necessitasse di proposte coraggiose e innovative, e che almeno si potesse provare ad uscire da quella grande emergenza con l'idea di non tornare semplicemente al passato. L'accesa discussione tra le forze politiche per eliminare il voto numerico nella scuola primaria e sostituirla con un giudizio descrittivo faceva parte di quella riflessione, con la consapevolezza quindi che la pandemia e, ad esempio, la scelta obbligata della didattica a distanza avessero fatto emergere ancora di più le contraddizioni della scuola italiana. Si cominciava a vedere assai meglio quello quello che alcuni di noi dicevano da tempo: l'istruzione pubblica, quel grande pilastro democratico attorno al quale si era costruita buona parte dell'idea dell'emancipazione sociale, innervando davvero i valori più alti contenuti nella Costituzione repubblicana, non era certo esente dal rischio di una torsione classista. La pandemia stava soltanto accentuando e rendendo più evidente quello che esisteva già, e che, attraverso troppe riforme sbagliate, stava minando alla base quella colonna portante che i Padri costituenti vollero fondare sull'inclusione e sulla democrazia. Quella del giudizio descrittivo era una piccola grande rivoluzione, una vera e propria innovazione contro la tirannia del voto, perché i bambini non possono essere considerati dei numeri; perché un 4 non può essere un macigno pesante da comprendere, mentre una valutazione complessiva prende in considerazione molto meglio le caratteristiche di un bambino; perché un voto numerico spesso significa giudicare non quel giovanissimo studente, ma il livello di istruzione della sua famiglia di origine. Oggi il Governo Meloni rivela, con questa scelta, con la pessima idea di tornare al passato, il suo carattere profondamente classista. Senza alcun monitoraggio, snobbando totalmente gli appelli dei pedagogisti e delle associazioni, riporta indietro l'orologio, come se si volesse recuperare l'autorevolezza perduta della scuola italiana attraverso l'autoritarismo; come se il modello a cui si guarda fosse quello opposto rispetto al ruolo emancipativo e trasformativo dei percorsi formativi, che invece necessiterebbero di tutt'altro: innanzitutto di risorse più adeguate per tutto il personale della scuola, a partire dal sostegno, o ancora di ridurre il numero degli studenti per classe, condizione essenziale - questa sì - per una scuola capace di rimuovere o almeno contrastare la disuguaglianza sociale. Voi avete scelto di non ascoltare la scuola e quell'esercito di maestre e maestri che ogni giorno svolgono un lavoro straordinario e del tutto malpagato, nonostante le enormi responsabilità sociali, culturali e formative a cui adempiono. È davvero insopportabile e contraddittorio che parliate ancora di merito, senza garantire una uguaglianza di opportunità. Come si fa a non capire che non c'è merito, se una gara è truccata, - per fare cento metri - qualcuno parte da zero e qualcun altro parte da cinquanta? Qual è il merito di cui parlate, se non sono garantite le pari condizioni di partenza? Non servono certo graduatorie o classifiche per le bambine e per i bambini. Serve, piuttosto, migliorare le informazioni descrittive, che aiutano gli allievi a conoscere se stessi e a essere orientati a dirigere la propria attività futura. L'insegnante ha con loro una relazione educativa. Non è un giudice ed è opportuno che sia il più possibile lontano da questo ruolo. La scuola può sollecitare a conoscere e a studiare, se aiuta a crescere senza mortificare, giudicare ed intimorire fin da piccoli, con il bollo di un voto numerico che esprime un valore sulla persona. Il voto, in realtà, è soltanto è soltanto una delle possibili scelte comunicative della valutazione e non è certo la scelta più efficiente. Se la finalità è quella di migliorare l'apprendimento, attribuire al voto la funzione di stimolo e di fine dell'apprendimento, è uno dei più gravi errori che si possa commettere, dato che spesso, peraltro - come è noto - porta a sviluppare atteggiamenti negativi verso la scuola e, più in generale, verso lo studio. Confondere, quindi, la valutazione col voto e attribuire ad esso la funzione di stimolo dell'apprendimento significa davvero non avere alcuna cognizione della complessità della questione. Agli inizi della grande scolarizzazione del mondo contemporaneo ci fu una fortissima richiesta di quelle competenze di base che, all'epoca, si riassumevano nella formula: leggere, scrivere e far di conto. conto. Rispetto a questo traguardo, anche i Paesi più avanzati, ancora una volta e anche in questo caso, come la pandemia ha drammaticamente disvelato, stanno verificando e soprattutto stanno vivendo un vero e proprio analfabetismo di ritorno. però, di confrontarsi con questo grande tema, con questa grande questione, di contrastarla in qualche modo, il Governo sceglie di ritornare indietro, di ritornare a una visione tremendamente classista, che ripete retoricamente la parola merito, tradendo però, nei fatti, il richiamo agli studenti meritevoli che esiste nella Costituzione italiana, la quale si poneva invece l'obiettivo, giustamente, di rimuovere gli ostacoli legati alle diverse condizioni di partenza. Io esprimo la nostra totale contrarietà a questo provvedimento, miope, autoritario e classista, che genererà demotivazione e paura di sbagliare, il contrario, cioè, della fiducia e della motivazione a migliorare che dovrebbero invece rappresentare i valori di fondo della scuola italiana. Con questo provvedimento, con la cultura politica che lo ispira, avete dimostrato, ancora una volta, di essere portatori di un pensiero profondamente reazionario. Il mondo, però, va avanti, nonostante voi proviate a riportare indietro le lancette della storia, e sarà sempre più forte di ogni nostalgia.

relativamente alla scuola secondaria di primo grado, cioè la scuola media che - come sappiamo tutti - costituisce un passaggio importante nella crescita e per la crescita dei nostri ragazzi. Infatti, lì si passa proprio dall'infanzia all'adolescenza. Siamo quindi intervenuti su questo. Per quanto riguarda, in particolar modo,

un ritorno al passato e - mi sia consentito un giudizio personale - secondo me stiamo facendo bene nel ritornare a certe sane abitudini del passato, perché un tempo, anche nella mia scuola, c'era il giudizio con

volta. Il giudizio in decimi, se viene espresso su una base di criteri oggettivi, rappresenta un elemento di chiarezza e di valutazione. Lo spazio del giudizio, quindi, è più ampio ed è anche maggiormente comprensibile. Positiva, oltre a queste, è anche la disposizione che l'alunno non venga ammesso alla classe successiva quando il giudizio sul comportamento sia inferiore al 6,

il giudizio complessivo a riflessioni ed elaborati dello studente che abbia preso un 6 durante il colloquio finale. Così come è certamente da considerare con favore il fatto

che la scuola, in generale, deve recuperare la propria autorevolezza. La scuola, lo voglio ricordare, è un'istituzione fondamentale del nostro Paese e tale deve essere considerata dai ragazzi. È quindi anche una

tempo, quando si veniva rimproverati a scuola e si tornava a casa, si prendevano gli altri rimproveri successivi, mentre oggi accade forse qualcosa di diverso, perché quando si torna a casa i genitori si arrabbiano perché c'è stato un comportamento diverso dell'insegnante. Questo, secondo me, non va bene. Il rispetto

ore e momenti della giornata importanti, che vanno condivisi con la famiglia. Allo stesso tempo, bisogna cercare di prevenire il disagio giovanile, che spesso è generato anche da situazioni familiari. Ecco quindi che ogni attività dei giovani, oltre il tempo passato tra i banchi scolastici (come sport, musica, arte

successive al percorso scolastico, possono essere importanti per coinvolgere il ragazzo e far maturare un comportamento sicuramente diverso e più proficuo. Dall'intera giornata del ragazzo deve nascere il basilare rispetto verso chi ci lavora e i docenti non possono diventare parafulmine di carenze educative. Il giudizio con voti numerici deve essere quindi basato su parametri oggettivi e deve tener conto della realtà in cui vivono i ragazzi. Per tali motivi, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. rappresentanti del Governo, fin dal principio il MoVimento 5 Stelle ha mosso ed evidenziato forti criticità sul provvedimento in oggetto, principalmente per tre ordini di ragioni. In primo luogo, per un'impostazione di fondo meramente punitiva e sanzionatoria. per le vaghe e indeterminate attività di cittadinanza solidale cui gli studenti dovrebbero sottoporsi e partecipare in seguito alla sospensione e al conseguente allontanamento dall'attività didattica. Infine, per la totale mancanza di una *pars construens*, ovvero di una parte costruttiva che possa bilanciare la parte sanzionatoria. Comminare una pena o una sanzione può essere più o meno opportuno, a seconda dei casi; tuttavia, non porta a nulla e, anzi, può addirittura avere effetti deleteri se non vi è un orizzonte capace di dare un senso e un valore a quel percorso: il senso di tramutare l'isolamento in socialità, la difficoltà in relazione o, ancora, di trasformare una cattiva condotta in una reale comprensione di un errore. In buona sostanza, se si vuole davvero ripristinare la cultura del rispetto, affermare l'autorevolezza dei docenti, nonché rimettere al centro il principio della responsabilità (sono tutte espressioni utilizzate nel testo che ci apprestiamo a votare oggi), restituendo piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, non basta prevedere il ricorso a un impiego temporaneo nei lavori socialmente utili. Ci troviamo quindi a discutere, per l'ennesima volta, di un provvedimento che riguarda la scuola pubblica italiana e che si concentra solo sul lato repressivo, senza alcun tipo di investimento reale nella parte preventiva. È il segno della scelta scientifica di questo Governo di utilizzare la scuola pubblica come strumento di propaganda e non come oggetto di investimento per una reale emancipazione dei nostri ragazzi e del Paese in generale. Concordiamo assolutamente sulla necessità di rafforzare una cultura del rispetto nei confronti dei docenti e del personale scolastico. I docenti vanno valorizzati sul piano professionale, economico e sociale e vanno evidentemente protetti da episodi di violenza fisica, psicologica o di qualunque altra natura. Tuttavia, il punto è come attuare questa valorizzazione e questa tutela. Davvero pensate che per fare questo sia sufficiente reintrodurre i giudizi e puntare solo su sospensioni e bocciature? Il rispetto è, prima di ogni altra cosa, un sinonimo di fiducia, che è esattamente tutto quello che state facendo mancare alla comunità scolastica e all'istituzione della scuola nel suo complesso. Va detto con onestà e chiarezza che, senza investimenti, qualsiasi intervento nella scuola sarà vano, sarà uno spot, sarà appunto propaganda. Il mondo della scuola ha dato una grande prova di resistenza e di reazione nel periodo Covid. Ma perché questo sia potuto avvenire è stato necessario sostenerla. Sapete a quanto è ammontato l'investimento nel comparto scolastico del Governo Conte per far fronte alla pandemia in un anno soltanto? 10 miliardi di euro. Sapete invece a quanto ammonta l'investimento di questo Governo per ogni scuola, con il soltanto sbandierato inserimento dell'educazione civica nelle scuole? Sette euro. Provate a trovare le differenze tra questi due investimenti, tra queste due cifre. *(Applausi)*. Purtroppo, la propaganda di questo Governo si può comprendere semplicemente unendo i pezzi di un *puzzle* che è decisamente preoccupante. Pensiamo agli accorpamenti selvaggi che avete messo in atto sotto il nome di dimensionamento, andando a indebolire i territori più fragili come quelli del Sud e delle aree interne del Paese che già soffrono di più la dispersione scolastica. dispersione scolastica. Quest'ultima è una vera e propria emergenza alla quale destinare attenzione e risorse. Se a questo aggiungiamo la distruzione del sistema scolastico nazionale con lo spacca-Italia, l'umiliazione come strumento educativo - questo dice il Ministro - il flop totale del liceo del *made in Italy*, allora il quadro diventa davvero terrificante. E che dire poi del rapporto di questo Governo con gli studenti di origine non italiana e con le loro famiglie? Ma davvero pensate che, con tutti i problemi che ha la scuola italiana, ci sia bisogno di un provvedimento per impedire la chiusura di un solo giorno di scuola per una festività religiosa? Non pensate che le scuole siano abbastanza sagge da capire come comportarsi nei vari singoli casi in base alle singole esigenze e caratteristiche? Ma poi, non eravate quelli a favore dell'autonomia? Di quale autonomia parlate, se poi, quando una decisione autonoma non vi piace, fate di tutto per modificarla attraverso atti decisi a livello centrale? Se fate così, infatti, la vostra cifra - permettetemi - non è quella dell'autonomia ma è quella dell'ipocrisia che è una cosa leggermente diversa. La propaganda di questo Governo sulla scuola è iniziata, lo dobbiamo dire, fin da subito, inserendo la parola merito nella dicitura del Ministero. Il che, se realmente applicato, sarebbe assolutamente e chiaramente condivisibile, ci mancherebbe, se non fosse però che poi, nelle tante nomine che avete fatto e state facendo nei vari settori, ed in particolare in quello culturale, la sensazione mia, ma sicuramente sarà sbagliata, è che per voi contino di più del merito la tessera di partito, la parentela e l'amicizia. Il merito lo avete messo soltanto nel titolo di un Ministero ma si è fermato a questo. Purtroppo, è l'intero impianto repressivo su cui si fonda la vostra politica la cosa più preoccupante in assoluto. State costruendo un mondo nel quale i giovani che non rispondono al vostro modello di società e che esprimono dissenso, dentro le scuole vanno incontro soltanto a sospensioni e bocciature senza nessun investimento nel sostegno, mentre fuori dalle scuole vanno incontro, più tristemente, anche alle manganellate. Se esiste una speranza di sovvertire questo modello di società che sta tradendo la scuola pubblica, la sanità pubblica, la giustizia e anche la libera informazione, bene, quella speranza sta proprio nei giovani che scendono in piazza. La pura repressione è un tradimento verso un'intera generazione. La pandemia ci ha restituito una società in cui la questione del disagio giovanile dovrebbe essere centrale e ci dovrebbe preoccupare tutti, mentre qui si continuano a fare dichiarazioni strampalate, provvedimenti di pura propaganda come questo. Il clima aggressivo che i ragazzi respirano nell'ambito dei *social* si riversa poi dentro e fuori le scuole. Queste ragazze e questi ragazzi, secondo voi, hanno bisogno soltanto di punizioni o forse hanno bisogno anche di supporto, di sostegno e di comprensione? Perché non mettete lo stesso impegno che mettete su provvedimenti esclusivamente repressivi come questo, anche su misure come il supporto psicologico o l'educazione affettiva e sessuale? Su questo vorrei dire che il MoVimento 5 Stelle ha presentato molti emendamenti per riempire il vuoto che c'è in questo testo. Abbiamo provato ad essere propositivi come al solito, abbiamo parlato di inserimento dello psicologo all'interno del sistema scolastico, di implementare l'attività sportiva, di implementare l'attività musicale. A tutto questo avete detto no. Non è possibile credere che pensiate davvero che il sistema scolastico si possa migliorare attraverso un progetto di scuola autoritaria, in cui lo strumento di contrasto principale diventa il voto in condotta o comunque la valutazione sintetica, piuttosto che quella descrittiva. In conclusione, il ministro Valditara si presentò ad inizio legislatura, dicendo che l'umiliazione è un fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità. Ecco, questa affermazione ha avuto un merito, cioè quello di farci capire subito in quali mani fossimo finiti e a più di un anno di distanza da quella frase, infelice, ci sentiamo di dire una cosa al Ministro. Se l'obiettivo di quella frase era dire che i ragazzi vanno educati con l'umiliazione, dobbiamo rispondergli con fermezza che sta sbagliando tutto, ma se il senso di quella frase era annunciare l'obiettivo di questo Governo di umiliare la scuola pubblica, allora state andando veramente alla grande. *(Applausi)*. Signora Presidente, per tutti i motivi fin qui esposti, annuncio il voto contrario del MoVimento 5 Stelle.

il disegno di legge che giunge oggi in discussione in Aula nella sua semplicità è particolarmente importante. Esso, infatti, è un tassello indispensabile di quel complessivo disegno di riorganizzazione e riqualificazione della scuola italiana a cui sta lavorando, sin dal suo insediamento, il Governo e il ministro dell'istruzione e del merito Valditara. Gli studenti rappresentano, insieme a docenti e genitori, uno dei tre assi portanti attorno a cui ruota l'istituzione scolastica; si può dire che essi siano il centro di tutto il processo formativo. Quel che però si è dimenticato per troppi anni è che la formazione è composta da due elementi che vanno assolutamente tenuti insieme e che sono di pari dignità: l'istruzione e l'educazione. Detto altrimenti, la scuola non deve limitarsi a trasmettere agli allievi conoscenze e metodi di apprendimento, ma deve porre una particolare attenzione anche ai loro comportamenti. Il suo fine è infatti anche quello di aiutarli a forgiare la propria personalità e il proprio carattere in previsione del loro ingresso in società come cittadini liberi e consapevoli. Non si è trattato di una dimenticanza casuale: la sottovalutazione dell'educazione è il portato diretto del predominio, dopo il Sessantotto, di ideologie politiche pedagogiche basate su una falsa idea di democrazia e di uguaglianza. In base ai loro dettami si è infatti finito per porre sullo stesso piano insegnanti e allievi, contestando quel principio di autorità che è fatto di rispetto dei ruoli e delle gerarchie e che è assolutamente essenziale per la buona riuscita del processo formativo. Alcuni studenti si sono quindi sentiti liberi di comportarsi come meglio credevano, in modo del tutto irresponsabile, in quanto l'idea stessa di una valutazione del loro comportamento da parte degli insegnanti è stata messa in discussione. Quanto ai docenti, persa ogni autorevolezza, è stato impedito loro di fare il proprio mestiere, li si è relegati al ruolo di consiglieri alla pari degli studenti, nel migliore dei casi, e di capro espiatorio per i loro *deficit* formativi nel peggiore. Gli episodi di violenza e bullismo di cui sono state piene le cronache dell'ultimo periodo possono perciò considerarsi la conseguenza di una situazione di fatto che è andata inesorabilmente deteriorandosi con il passare degli anni. Alla luce di questa situazione si è perciò reso necessario intervenire per ripristinare nelle aule scolastiche la cultura del rispetto attraverso la valorizzazione a più livelli del voto di comportamento nelle scuole di ogni ordine e grado. Ciò nella consapevolezza che ha sempre accompagnato la cultura classica occidentale nel suo sviluppo storico che educazione ed istruzione non possono andare disgiunte, ma sono i due poli di un unico processo. La novità di questo disegno di legge è che esso supera il precedente approccio punitivo e sanzionatorio, favorendo meccanismi di recupero che coinvolgono lo studente in attività didattiche, oppure, nei casi più gravi di allontanamento dalla scuola, in attività sociali presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche. Si cerca di favorire altresì i processi di riflessione critica e autovalutazione degli studenti sul proprio operato. Contestualmente, per favorire l'indispensabile partecipazione delle famiglie nel processo formativo, il disegno di legge affronta una criticità presente nell'attuale sistema di valutazione delle scuole primarie. In esse il giudizio dato in pagella, essendo molto analitico e specialistico, non rende infatti facilmente e immediatamente visibile ai genitori il livello di apprendimento che i loro figli hanno raggiunto. Alla valutazione analitica, che resta e non è stata soppressa, al contrario di quanto i *media* hanno spesso erroneamente detto, si è perciò ritenuto opportuno affiancare una valutazione sintetica di facile leggibilità. può dirsi che i provvedimenti presi si propongano di ristabilire un clima di serenità e collaborazione nelle scuole: senza questo clima, la scuola italiana non può lavorare unita per affrontare le enormi sfide che l'attendono. Su di esse si giocherà non solo il suo futuro, ma anche quello del nostro Paese. È perciò necessario non abbandonare le nuove generazioni a se stesse. A nome della Lega, quindi, annuncio un convinto voto favorevole al provvedimento in

Mi sono chiesta, leggendo questo disegno di legge, se siamo ancora capaci di sognare le bambine e i bambini e le ragazze e i ragazzi che vivono nel nostro Paese. Noi, un Paese che invecchia, come ci dicono tutte le statistiche sulla denatalità, per motivi vari - fatemelo dire - a cominciare da uno scarto enorme tra figli desiderati e realizzati, siamo dunque un Paese ingiusto, soprattutto con le donne. Eppure, anche nel dibattito di ieri, ho sentito ancora qualcuno parlare di cattive letture e di narrazione sbagliata sulla maternità altro sostenere che bisogna indottrinare e omettere qualche associazione pro-vita nei consultori: altro che narrazione tossica, il 20 per cento delle madri lascia il lavoro dopo il primo figlio! Oltre al danno, la beffa: nessun rispetto per le scelte di maternità o di non avere figli e non venite a chiederci su questo dove eravamo, perché avevamo cominciato con un assegno universale, obiettivi di occupazione femminile, parità di genere, servizi educativi da nel PNRR, che voi avete completamente stravolto. *(Applausi)*. Ebbene, questo Paese anziano come guarda alle giovani generazioni? Come vuole educarle?

e che quindi vadano puniti: persino i più piccoli, quelli della primaria, si discute se possano essere insufficienti o gravemente insufficienti. Si tratta dunque di una generazione scarsa non nel rendimento, ma nel senso che sono pochi e, nonostante questo, invece di fare per loro classi più agevoli - come ha ricordato prima un mio collega - e meno numerose, scegliamo accorpamento e dimensionamento. È una generazione scarsa,

una risorsa scarsa, che decidiamo anche di selezionare, visto che parliamo di tetti, invece di cercare di capire come trattenerla quanto più possibile in questo luogo di educazione alla cittadinanza (organo costituzionale, come diceva Calamandrei). Trattenere, appassionare, coinvolgere: sembra proprio che invece dei più giovani sappiamo vedere solo gli sbagli, mettendo insieme occupazioni, episodi di violenza, disagio sociale e aggressività; emergenza-violenza, insomma, senza provare a capire cosa non funzioni, cosa abbia procurato il Covid, quale patto si sia rotto. Qualcosa si è rotto, infatti, anche nel rapporto con le famiglie e qualcosa si è rotto tra i ragazzi, perché la violenza spesso la fanno anche a se stessi *(Applausi)*, tra autolesionismo e disturbi alimentari. Qualcosa si è rotto davvero.

con la storia del '68 e del 6 politico? Dopo quarant'anni di rivoluzione neoconservatrice e di liberismo, in cui competizione e individualismo hanno avuto la meglio, veramente parliamo ancora di questo? Davvero volete accusarci di pensare che vada tutto bene, che non ci siano problemi nella scuola italiana e che non ci sia un problema di riconoscimento di autorevolezza? Altrimenti noi siamo i secchioni, quelli che giudicano. Francamente, a sentir parlare di Gattopardo e di Time Square, un po' di giudizio ci verrebbe da darlo. Ma sinceramente stiamo parlando di una cosa importante e delicata come la valutazione. Riusciamo a uscire da questa discussione ideologica e stereotipata? Noi l'abbiamo letto sul serio e, quando avete citato grandi pedagogiste, sia gli emendamenti che gli articoli li abbiamo anche votati, perché abbiamo guardato al merito di questo disegno di legge. Certo che vediamo i problemi; abbiamo anche detto di voler investire di più sulla comunità educante, indicando, negli emendamenti, le figure che possono sostenerla e arricchirla. In gioco c'è che tipo di scuola vogliamo e che cos'è l'autorevolezza, che è anche data dal riconoscimento sociale e salariale del lavoro dell'insegnante. Però qui la china scelta è quella dell'autoritarismo. L'insegnante tornerebbe a fare la sua parte nel saper punire;

È oggettivo questo potere, va maneggiato con cura, può essere inteso come una funzione sanzionatrice, selettiva e di controllo, oppure come uno strumento di promozione della persona, con una funzione educativa e di rinforzo positivo: la scuola che rimuove gli ostacoli, la scuola costituzionale che rimuove gli ostacoli. Può essere un giudizio secco oppure un processo, una mossa riflessiva per chi è giudicato e per chi giudica, di comprensione su quale strada intraprendere con quel percorso didattico. Il voto è una sintesi ordinale, stila graduatorie, innesca competizioni e paragoni, tende a riprodurre e a legittimare le diseguaglianze di partenza. La competizione, questo è stato il *mantra* di questi anni, che ammazza il gruppo classe, lo studio condiviso, il rapporto tra pari. Questi sono i problemi che abbiamo visto nelle scuole. Questo disegno di legge era stato pensato in origine per disciplinare il voto in condotta, entrando nei dettagli, volendo spiegare agli insegnanti esattamente come devono fare, anche se poi le fattispecie che determinano la non ammissione rimangono ampie e ambigue. Nessuna intenzione di recupero, ma solo rigidità; di fatto, una messa in discussione della valutazione collegiale. Esso poi modifica anche lo statuto degli studenti e delle studentesse; i principi generali, ha detto la relatrice. Ma quei principi generali vanno condivisi con gli studenti e le studentesse. *(Applausi)*. Quel testo, all'articolo 4, parla di disciplina e dice chiaramente che nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni; nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Qui invece siamo proprio alla controrivoluzione, alla reazione; qui si instaura un automatismo che porta al non passaggio alla classe successiva. Su un provvedimento siffatto è arrivato l'emendamento che introduce il giudizio sintetico nella primaria, cassando quell'ordinanza del 2020 che - come è stato ricordato - è stata emanata in pieno Covid, in un momento in cui la scuola soffriva, in cui aveva la didattica a distanza e in cui sono esplose le criticità, i problemi e le diseguaglianze. Su quella sperimentazione è stata fatta formazione; la scuola richiedeva da tempo, dal 2008 (quando erano stati cancellati), che si tornasse al giudizio descrittivo. Nel 2020 si avvia quindi finalmente una riforma che riporta la valutazione descrittiva; tante associazioni hanno chiesto di non tornare indietro e, soprattutto, di non farlo senza aver fatto una valutazione e aver verificato l'efficacia, di non interrompere, a ogni Governo che arriva, un percorso che la scuola ha iniziato. Questo cambiamento della valutazione riguarda infatti la didattica. Come si valuta è fortemente legato alla didattica. Se l'attività è concepita solo come spiegazione, interrogazione, valutazione o se invece la valutazione non orienta un processo, ma non per rendicontare e classificare. È questo il motivo per cui noi siamo critici rispetto a questo disegno di voto. Concepire il voto come modalità prevalente nella comunicazione del processo valutativo è coerente con la scelta di classificare e riprodurre le diseguaglianze. E qui torniamo al sogno - concludo, Presidente - e a come guardiamo alle bambine e ai bambini, a come vogliamo sognarli. Una didattica che considera elementi fondamentali della propria azione il coinvolgimento attivo e la condivisione del potere valutativo. Non si educa infatti alla democrazia sviluppando sudditanza, ma promuovendo partecipazione attiva e facendosi carico delle responsabilità che tale partecipazione comporta, a cominciare dal lavoro sugli errori commessi, senza dimenticare lo stress e il terrore di sbagliare di tanti ragazze e ragazzi che trasmettono avversione verso l'apprendimento. Avete scelto la strada sbagliata della punizione e del controllo anche degli insegnanti. Per questi motivi, dichiaro il voto contrario del Partito Democratico.

di introdurre strumenti punitivi nei confronti delle studentesse e degli studenti italiani, né tantomeno bacchettate sulle mani o altre forme che sembra siano state evocate evocate in molti degli interventi dell'opposizione. Semmai, quello che rilevo è che ci sono molte forze politiche che hanno fatto parte di Governi sui quali è stata costruita la scuola che abbiamo oggi e che non hanno espresso nemmeno una parola riconoscendo le proprie responsabilità sui tanti errori - in qualche caso orrori - presenti nelle scuole italiane. Il fatto di non riconoscersi delle responsabilità è proprio il modo col quale loro interpretano anche l'educazione che dovremmo dare ai nostri figli, ai bambini, agli adolescenti e agli studenti italiani, cioè quello di non assumersi le responsabilità. Quello della responsabilità è un tema da cui evidentemente la politica, soprattutto quella che sta dall'altra parte dell'Emiciclo, rifugge.

intellettuale che certamente non è ascrivibile a questa parte politica, ossia Galli della Loggia, qualche tempo fa ha fatto una richiesta alla politica perché si reintroduca il predellino all'interno delle classi per mettere in condizione gli insegnanti di avere, da un lato, la possibilità di controllare meglio quello che succede nella classe, e dall'altro lato di vedersi riconosciuta quell'autorevolezza *(Applausi)* che purtroppo invece troppo spesso non viene loro riconosciuta nelle classi italiane. Gli obiettivi che si pone questa legge sono quelli di migliorare il rapporto tra gli studenti, il personale docente e il personale amministrativo delle scuole. Migliorare i rapporti,

che molto spesso questo rapporto di civiltà e di rispetto tra studenti e studenti, tra studenti e insegnanti, tra studenti e personale amministrativo, purtroppo nella scuola italiana si è perso. Riportare la cultura del rispetto degli ambienti scolastici è un obiettivo che si pone questo provvedimento, così come quello di far comprendere agli studenti l'importanza di un comportamento responsabile e rispettoso verso gli altri. Scandisco ancora la parola "responsabile". La valutazione del comportamento non deve essere vista come un voto di serie B rispetto alle materie curricolari. Nessuno vuole condizionare il profitto rispetto al comportamento, però è uno dei parametri più importanti nella valutazione complessiva che, come istituzione scolastica, possiamo dare dello studente. Una valutazione che non deve e non può tenere conto solo del rendimento nelle singole materie, ma anche dell'approccio generale dello studente nell'ambiente scolastico e nelle relazioni con gli altri.

riveste questo tipo di funzione: quella formativa. Quindi, la valutazione del comportamento non deve avere una funzione meramente punitiva, ovviamente, ma deve servire innanzitutto allo studente, per capire se il suo comportamento non è consono all'ambiente scolastico e offrirgli, in questo modo, anche la possibilità di migliorare. Ecco perché riteniamo particolarmente importante coinvolgere gli studenti che dovessero ottenere una valutazione intermedia insufficiente in attività quali quella della cittadinanza attiva e solidale, come richiesto dalla disposizione introdotta dalla Commissione. La stessa cosa vale per gli studenti che ricevono il provvedimento di allontanamento dalla scuola. La sospensione è molto più utile se accompagnata da un'attività di riflessione e di servizio solidale presso strutture convenzionate, un'attività che sicuramente può stimolare lo studente ad approfondire le motivazioni del provvedimento disciplinare che ha ricevuto e a comprendere la gravità delle proprie azioni. Io capisco, sì, che che debba esserci la misericordia, la comprensione, e che la ricerca di tutti noi debba essere quella di mettere tutti nella condizione di procedere sui giusti binari, ma dobbiamo anche educare al senso della giustizia. *(Applausi)*. Il senso della giustizia, come diceva una pedagoga che ho conosciuto, che era mia nonna, è che, quando fai le cose giuste, ricevi un premio, ma se sbagli, devi assumerti la responsabilità dell'errore e devi anche ricevere un elemento punitivo. Questo non significa trasformare la scuola in un ambiente autoritario, come ho sentito dire, ma trasformare la scuola in un ambiente formativo, non autoritario. Anche la sospensione del giudizio per gli studenti ammessi agli scrutini finali con la valutazione di sei decimi è una novità molto positiva: non comporta la bocciatura diretta, ma richiede uno sforzo in più dello studente in termini di approfondimento e di elaborazione per ottenere la piena ammissione alla classe successiva. successiva. Anche in questo caso, la volontà, la finalità, non è certo quella di punire, ma di dare l'opportunità a tutti di imparare dai propri errori e diventare più responsabili. Se, a fronte di queste misure, il comportamento dovesse essere comunque ritenuto insufficiente da parte del consiglio di classe, allora sì, certo, lo studente dovrebbe necessariamente ripetere l'anno, come come purtroppo è accaduto a generazioni di studenti che, grazie a quegli errori e a quegli anni persi, hanno conquistato, invece, valori importanti da spendere nella loro vita.

sintetici, non numerici. E vi è una differenza, non solo lessicale, ma importante anche dal punto di vista del contenuto. è stato il voto all'unanimità sull'emendamento presentato dal collega di Fratelli d'Italia, Paolo Marcheschi, che estende l'inserimento del metodo Montessori, per chi vorrà adottarlo, alle scuole primarie. Ovviamente, non si obbliga alcuno ad adottare questo sistema, ma si mette in condizione, chi ritiene utile adottarlo, di poterlo fare. Per noi è fondamentale che i reati commessi contro il personale scolastico non siano puniti soltanto con il risarcimento dei danni alla singola persona offesa (perché anche questo è un caso che oggi si verifica) ma che si preveda anche un risarcimento alla scuola. Questo perché un comportamento violento e irrispettoso non è solo un danno alla persona, ma un danno grave all'intera comunità In conclusione, signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia, che voterà a favore di questo provvedimento, ritiene che anche la scuola debba fare la sua parte nel permettere ai ragazzi di sviluppare la propria coscienza, anche attraverso una necessaria assunzione di responsabilità da parte di questi, rispetto innanzitutto a se stessi e poi, di conseguenza, rispetto agli altri. I comportamenti di oggi in ambito scolastico riflettere, e spesso drammaticamente riflettono, i comportamenti di domani nel mondo del lavoro e, più in generale, nelle complesse relazioni sociali. Il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore del

di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi didattici differenziati». *(Segue la

del responsabile del coordinamento unitario in difesa del patrimonio bufalino, Gianni Fabbris, insieme ad un rappresentante campano Adriano Noviello e a Sebastiano Lombardo della Sicilia. In realtà loro sono i rappresentanti degli allevatori bufalini di quattro regioni

si sono interessati anche i colleghi della maggioranza dei territori coinvolti. Quindi, chiediamo che si possa intervenire a difesa degli allevatori che ricordano gli ultimi casi di brucellosi, prendendo ad esempio il Comune di Castel Volturno, in Campania, in provincia di Caserta, dove solo negli ultimi due mesi ci sono stati 11 focolai, 11 casi avvenuti in altrettante aziende che hanno comunque subito il piano di eradicamento previsto dalla Regione Campania.

La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito di posticipare alla seduta di martedì 23 aprile alle ore 13,30 l'inizio della discussione del decreto-legge in materia di ulteriori disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di permettere alle Commissioni bilancio congiunte di Camera e Senato di svolgere le audizioni sul Documento di economia e finanza 2024. La seduta di lunedì 22, pertanto, non avrà luogo. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia sul decreto-legge, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che la chiama avrà inizio alle ore 18,30 della stessa giornata di martedì. Resta confermata per la seduta di mercoledì 24 la discussione del Documento di economia e finanza. Il sindacato ispettivo di domani non avrà luogo. Pertanto la seduta di domani avrà inizio alle ore 15 per lo svolgimento del *question time*. L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 30 aprile alle ore 10 con la discussione di ratifiche di accordi internazionali. Resta confermata la convocazione del Parlamento in seduta comune martedì 23, alle ore 12,30 ore 12,30 per la terza votazione concernente l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli senatori.

Signor Presidente, in merito ai fatti che si sono verificati all'Università «La Sapienza», stiamo vivendo una fase estremamente preoccupante. sinceramente che non riesco a comprendere come possa accadere che gli studenti universitari vadano ad impedire

tutta la nostra solidarietà e mostrarla a quel dirigente della Polizia di Stato che è stato letteralmente malmenato e preso a pugni, perché questo non è manifestare, come qualcuno ha dichiarato sulla stampa, su alcuna stampa patinata. Questo vuol dire adottare degli atti assolutamente criminali.

Andiamo ad accettare questi atti di antisemitismo oggi, come quelli che si sono verificati nei riguardi di Parenzo, a cui è stato impedito di parlare qualche giorno fa, o così com'è accaduto - lo ricordo - il 2008 al Santo Padre, Papa Benedetto XVI? Tutto ciò è assolutamente inaccettabile ed è per questo che richiamo veramente all'attenzione tutte le forze politiche, perché noi non possiamo accettare che si ricrei un certo clima, come purtroppo si sta verificando. Le parti politiche che non condannano fatti del genere si rendono responsabili del clima politico che si sta ingenerando tra i nostri giovani e che, purtroppo, non può che rievocarci pagine tristi, quale quella che è stata richiamata ieri nel momento commemorativo dal senatore Andrea De Priamo, rispetto ai fatti verificatisi nei confronti dei fratelli

Signor Presidente, il mio è un intervento per un pensiero commosso che voglio rivolgere a una persona, che purtroppo pochi giorni fa ci ha lasciati. Faccio riferimento a Giovanni Paolo Bernini, ex assessore a Parma,

ma soprattutto una persona che ha creduto fortemente nella necessità di far emergere la verità da una vicenda personale che lo ha visto coinvolto, purtroppo indagato e imputato, addirittura soggetto a misure cautelari, grande inchiesta che doveva far luce sui rapporti tra politica e criminalità organizzata in Emilia-Romagna; che lo ha visto appunto coinvolto, insieme a un'altra figura di secondo piano, sempre di Forza Italia, e poi completamente scagionato da ogni accusa. Di più:

quanto accaduto in quella storia. Giovanni Bernini in realtà lo vorrei ricordare per la grande umanità e il grande senso di altruismo che ha sempre avuto nei confronti di tutte le vittime della giustizia. Ha coadiuvato il sottoscritto nel corso della campagna referendaria sui referendum della giustizia di due anni fa e soprattutto non si è mai tirato indietro, anche attraverso opere monografiche che ha scritto sulla sua vicenda, dall'illustrare quanto la giustizia male amministrata possa essere un male per tutti i cittadini che, in maniera del tutto indifferente, si trovano coinvolti in un servizio che a volte non funziona per problemi legati all'incapacità o, peggio, alla collusione di alcuni che decidono di non essere veramente integerrimi quando ricoprono incarichi istituzionali pubblici. Giovanni Bernini era una persona splendida: ai suoi familiari vadano tutta la nostra commozione e il nostro ricordo. Giovanni Paolo, riposa in pace e sappi che hai tanti amici, che continueranno le battaglie sulla giustizia anche per te.

oggi: è mercoledì e oggi pomeriggio non abbiamo lavori e, quindi, non avremo provvedimenti da votare; già la scorsa settimana l'ultimo provvedimento lo abbiamo concluso nel primo pomeriggio di mercoledì domani non c'è neanche il sindacato ispettivo, mentre la Presidente di turno la settimana scorsa mi ha rimproverato perché non ricordavo che ci fosse il sindacato ispettivo. Non è tanto una questione legata al Parlamento. La cosa che mi preoccupa è un tema tutto politico e cioè che, se le Camere non sono chiamate a deliberare su provvedimenti proposti dal Governo o dalla maggioranza, vuol dire che c'è un problema politico della maggioranza e del Governo di produrre atti legislativi per il governo del Paese. del Paese. Neanche dalle Commissioni arrivano provvedimenti, magari di iniziativa parlamentare, però proposti dalla maggioranza; quelli dell'opposizione non vengono calendarizzati; per quelli della maggioranza non ci sono voti; il Governo non ci porta niente, tranne voti di fiducia, come succederà la settimana prossima. Per me è un dato politico che va posto all'attenzione del Paese: questo Governo e questa maggioranza non stanno governando e non stanno producendo leggi, altrimenti non si spiega come mai noi, il mercoledì, alle ore 13, abbiamo concluso i lavori, perché non c'è altro. Non vengono calendarizzati provvedimenti: questo è un dato politico fondamentale.

e mi riservo di farlo ancora, se questo Governo non comincerà a fare cose, sulle quali probabilmente sarei in totale disaccordo. Una cosa però è giudicare un Governo e una maggioranza perché fanno cose che non piacciono, e magari non piacciono un pezzo dell'opinione pubblica. Altra cosa è dire all'opinione pubblica

del suo Gruppo. Tengo anche a sottolineare che le Commissioni sono riunite oggi e domani, come sappiamo, anche per la discussione del Documento di economia e finanza e di tanti altri provvedimenti.